Grazie, ha naturalmente un significato politico e parlamentare, ma anche un'attinenza al dettato dei nostri Regolamenti. È su questo insieme di fattori che vorrei richiamare l'attenzione della Presidenza del Senato e dell'Aula. Infatti, nella parte finale della seduta di stamattina la nostra Aula ha subito delle tensioni di particolare violenza che hanno influenzato e, in qualche momento, anche bloccato i lavori dell'Aula. Questo avveniva nella parte finale della discussione di un provvedimento in materia delicata: un provvedimento che ha visto impegnata l'Aula del Senato per molte sedute e ha visto anche fasi di vero e proprio ostruzionismo, che, nella parte finale, è a mio parere degenerato. Dico subito, per levare la questione dal campo, che non approvo minimamente l'irruzione del senatore Fasano del Gruppo PdL verso i banchi del Movimento 5 Stelle e ringrazio i senatori, anche del suo Gruppo, che l'hanno fermato. Ma la questione

abbiamo ascoltato le dichiarazioni di voto di tutti i Gruppi e, al termine di esse, praticamente tutti i senatori del Movimento 5 Stelle si sono iscritti a parlare per esprimere una dichiarazione in dissenso. questo ci interroghi su almeno due elementi delicati. si iscrive per dissentire dalla dichiarazione di voto del senatore che poco prima si è espresso a nome di tutto il Gruppo, è la maggioranza del Gruppo che ne di che dissenso parliamo se tutto il Gruppo ha una volontà diversa dal senatore che dal Gruppo è stato incaricato di parlare? *(Applausi dai Gruppi*

avete dei comportamenti parlamentari che non condivido; voi potete rispettare me se esprimo delle opinioni che non condividete. *(Applausi dai Gruppi* *PD e PdL).* Penso che ci sia qualcosa che non rispetta la logica, e la logica, anche in Parlamento, ha un senso.

che deve essere assegnato ad ogni singolo senatore che vuole esprimere un'opinione in dissenso dal proprio Gruppo. Ci sono state opinioni diverse: i senatori del Movimento 5 Stelle che sono intervenuti sostenevano di avere diritto a parlare per un certo tempo e il Presidente del Senato (chi in quel momento sedeva al banco della Presidenza del Senato) aveva una diversa opinione. Il nostro Regolamento prevede che in questi casi il Presidente del Senato prevalga con la sua volontà. Il nostro Regolamento prevede che la questione si chiuda con la decisione del Presidente del Senato. C'è ovviamente un rimedio C'è ovviamente un rimedio a cui molte volte nelle passate legislature si è fatto ricorso, ed è quello di porre la questione presso la Giunta per il Regolamento, perché c'è evidentemente una differenza di opinioni sull'interpretazione del Regolamento. Questa differenza non può essere sciolta in Aula, perché non è questa la sede, e va sciolta in Giunta. penso che male si faccia a trasformare una discussione regolamentare molto delicata, che investe diverse parti del nostro Regolamento, in una diciamolo pure - seduta degenerata, nella quale le urla superano gli argomenti, nella quale le interruzioni sono più frequenti della parola presa perché concessa dalla Presidenza,

Se un Gruppo politico (o soltanto un senatore) intende ostacolare l'approvazione di un provvedimento, anche di un provvedimento importante al quale la maggioranza tiene molto, se questo Gruppo (o questo senatore) si muove all'interno delle prescrizioni del Regolamento, devo dire che, anche non condividendo il suo comportamento, farò tutto quel che posso perché questo Gruppo possa svolgere la sua funzione, anche in forme ostruzionistiche. Ma se la protesta assume delle delle forme che mettono a repentaglio il sistema parlamentare, che possono essere interpretate o siano delle offese al sistema parlamentare e che abbiano come obiettivo il suo indebolimento, e tale è l'operazione di alzarsi in Aula e stracciare il volume che contiene il Regolamento e la Costituzione *(Applausi

Signora Presidente, mentre io chiedo alla Presidenza di proseguire in un'azione di rispetto di tutti i parlamentari a cominciare dalle opposizioni, nei loro comportamenti anche ostruzionistici, purché siano all'interno del Regolamento, contemporaneamente chiedo alla Presidenza di applicare in modo rigido il Regolamento nei confronti di quei parlamentari che non lo osservano e lo violano continuamente, perché questo non può essere tollerato dall'Aula. a chi dei nostri colleghi si alza ripetutamente ricordando

eletti per affrontare la crisi del nostro Paese e per difendere la Costituzione della Repubblica e non per stracciarla in Aula.

noi riteniamo che i Regolamenti abbiano una funzione: quella di essere depositari dei valori della nostra Costituzione,

valori sono centrati sull'accettazione del pluralismo, proprio perché il Parlamento deve essere il luogo in cui le persone si parlano, si ascoltano, recepiscono le indicazioni che provengono dall'altra parte (magari ascoltando non il collega di banco, ma tutti, soprattutto quando ci si rivolge direttamente all'altro), affinché - come lei ricordava, citando implicitamente Voltaire - venga rispettata la fondamentale libertà di ogni cittadino italiano di poter esprimere il suo pensiero nel rispetto che si deve a tutto ciò che è argomentazione, a tutto ciò che è razionalità, a tutto ciò che rimarca un pensiero che nasce da una riflessione che ha alle spalle un'esperienza di vita, che nasce da una crisi sociale e civile che noi siamo qui chiamati ad affrontare e risolvere. Mi si insegna, però, che l'Aula è il luogo in cui confluisce il lavoro delle Commissioni; pertanto, volendo avere memoria, domandiamoci anche perché si arrivi a questi atti che lei reputa di ostruzionismo

debba essere il più possibile avversato, reputandolo, nella sua complessità e nella sua genericità, addirittura peggiore della situazione che andrebbe a sanare. In Commissione - e qua le carte cantano - i nostri senatori hanno proposto un lavoro dialogante, un lavoro emendante, un lavoro volto a migliorare, non con la presunzione di avere tutte le verità in tasca, ma con l'umiltà di poter proporre nel dialogo delle vie per sanare delle situazioni che, a giudizio di tanti, e non soltanto del nostro Movimento, sono da sanare con immediatezza. In Commissione non c'è stata alcuna volontà di dialogo, come il sottoscritto ha rimarcato anche ieri pomeriggio al ministro Franceschini. Ora, a fronte di questo atteggiamento di assoluta chiusura, noi abbiamo reputato di

per quanto prevede l'articolo 109 del Regolamento, che leggo: «Uguale facoltà è riconosciuta ai senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal proprio Gruppo, purché il loro numero sia inferiore alla metà di quello degli appartenenti al Gruppo stesso». E le dico anche, collega Zanda, che, se il Regolamento del Senato fosse stato quello della Camera, probabilmente avremmo, come alla Camera, vissuto delle notti delle notti di discorsi, di interrogazioni, di interventi, perché ritenevamo che, per quello che ci viene concesso dal Regolamento... Ora, noi vorremmo che tutto questo avvenisse nel solco di un rispetto che tutti dobbiamo avere nei confronti di tutti. Ma molto spesso le maggioranze,

della mediazione, purché nasca da argomentazioni. Noi le argomentazioni le produciamo: siete voi che siete sordi, soprattutto in Commissione! Grazie,

ci siamo a volte anche scontrati dialetticamente e politicamente, ricorrendo spesso (non sempre) anche a misure ostruzionistiche. A volte è successo anche a me, signora Presidente, quando avevo l'onore di occupare quel banco, di dover garantire, come ho cercato di fare, a chi svolgeva un ruolo di opposizione l'esercizio dei propri diritti regolamentari, attraverso un ostruzionismo che si richiamasse al Regolamento, finalizzato a rallentare i lavori del Parlamento.

occorre sempre tenere a mente che esistono le regole della democrazia parlamentare, dove ci si confronta, ci si cerca di ascoltare quando poi vi sono dei momenti decisionali, scattano le regole della democrazia. La democrazia parlamentare prevede il voto. Lo prevede addirittura per per fissare l'esigenza o no di una prosecuzione dei lavori dell'Assemblea (pensate un po'), lo prevede nei momenti in cui in Aula si discute un argomento imprevisto e non vi è una condivisione dell'Assemblea. Tante volte il Presidente di turno mette ai voti quelle scelte sulle quali non vi è condivisione. La democrazia è questo: è il voto. So bene che alla Camera il diverso Regolamento avrebbe potuto consentire al Movimento 5 Stelle di impegnare quest'Aula per intere notti, come avete fatto con apprezzabile apprezzabile ed ammirevole spirito di sacrificio, perché l'Italia ha osservato impegnare l'Aula per intere notti: avete raggiunto un obiettivo - un obiettivo politico - ricorrendo alle vostre prerogative. Vorrei però ricordare soltanto due dati. Questo, colleghi, è un provvedimento delicato, su di esso vi siete battuti in Commissione per il recepimento delle vostre idee e non siete stati ascoltati: di questo prendiamo atto.

Vorrei quindi trarre da questa vicenda un elemento di grande chiarezza e di grande positività. Oggi quest'Aula, al di là della spiacevole vicenda che spero venga dimenticata, registra,

E lo dico con convinzione, perché quante volte da questi banchi si sono levate, manifestazioni di protesta nei confronti del Governo da parte delle opposizioni e a volte anche, più silenziosamente, da parte delle maggioranze che sostenevano i Governi e che subivano le questioni di fiducia? Questo non è successo, non si è verificato, ed è una dimostrazione di grande, grande, grande affermazione del ruolo del nostro Parlamento.

Quindi nessuna contestazione mi sento di muovere personalmente alle richieste di dichiarazione di voto in dissenso, nel rispetto del Regolamento. di Carte che contengono valori nei quali noi ci riconosciamo e di Regolamenti nei quali ci dobbiamo riconoscere fin quando non vengono cambiati, perché sono a garanzia di tutti, colleghi (oggi possono essere visti a nostra garanzia, un domani possono essere visti a vostra garanzia, la ruota della democrazia allora no: questi gesti vanno condannati, vanno dimenticati e non vanno ripetuti. E con questo concludo il mio intervento: ben venga il confronto in Commissione, ben venga il confronto in Aula, pronti ad ascoltare, pronti a confrontarci, ma facciamo in modo che

che non avrebbe consentito a nessuno di voi, ma a nessuno in quest'Aula di poter dire la propria sulle singole richieste emendative e, quindi, di poter esercitare quel mandato che ci hanno riconosciuto gli italiani quando ci hanno votato.

che l'ostruzionismo è una pratica seria, molto seria, e come tutte le cose serie noi, tutti insieme, nell'interesse di tutti, nell'interesse della democrazia, nell'interesse di quest'Assemblea,

E se mi permettete, anche il riferimento ai Padri della Patria, ai Padri costituenti, deve essere fatto con grande prudenza, con grande parsimonia,

di volerla violentare; ci richiamano ad una profonda differenza tra noi che rappresenteremmo la farsa e i Padri costituenti che rappresentano (come davvero rappresentano) la storia, la nostra fonte di ispirazione. Credo che questi paragoni impropri, queste esagerazioni, non siano utili a quello che vogliamo rappresentare in quest'Aula e a quello che vogliamo fare nel tentativo di adeguare le nostre istituzioni al bisogno di cambiamento che c'è nel Paese. Abbiamo bisogno di cambiare le fonti primarie del nostro diritto, le forme del nostro Governo per renderlo più adeguato ai cittadini, senza senza stravolgere la nostra democrazia, ma ricreando un rapporto di fiducia. Abbiamo bisogno che questo Parlamento produca efficacia. Talvolta, ad uno come me che non ci ha mai messo piede qui dentro fino al 15 marzo di quest'anno, sembra che sia una macchina molto efficiente, ma per nulla efficace, che costringe, ad esempio, il Governo a varare provvedimenti *omnibus* con 120 articoli che parlano di tutto e del contrario di tutto, perché il timore è di non riuscire a raggiungere l'obiettivo che una maggioranza che si forma nel Parlamento, organo sovrano della rappresentanza popolare, indica al Paese come una soluzione. Di qui i provvedimenti sconclusionati, e su questo concordo con il fatto che a volte siamo costretti a fare i conti con provvedimenti incoerenti tra di loro. Ma questo è figlio di Regolamenti parlamentari barocchi, di un modo di concepire la democrazia e anche il ruolo del parlamentare che non ha più nulla a che fare con l'aria che sta fuori dal palazzo, che non ha nulla neanche a che fare con quanto avviene nel resto d'Europa, nelle altre Assemblee, dove si lavora per sessioni, dove le discussioni generali al massimo sono momenti in cui un oratore interviene per due, tre, quattro, cinque minuti. Per sette Per sette anni sono intervenuto al Parlamento europeo su argomenti anche importanti, ma per non più di due o tre minuti. E non per questo mi sono mai sentito violentato nella mia rappresentatività democratica e popolare. Certo, vedere sventolare

perché l'esaltazione del nostro ruolo non sta nell'impedire a una maggioranza di governare, ma nel rivendicare lo spazio per poter affermare, dentro al palazzo e fuori dal palazzo, la nostra volontà. e credo che questo non sia stato minimamente negato al Movimento 5 Stelle. Credo che questo varrà anche nei prossimi appuntamenti, ma ritengo anche che dobbiamo davvero prenderlo come un impegno. Non sono la compressione della parola al singolo o la riduzione da dieci a tre minuti

ma sempre dentro una logica barocca. Io vi invito a non utilizzare questo strumento, vi invito a portare la battaglia di contenuto dentro le Commissioni,

perché questa è la logica con cui ci dobbiamo muovere. È un impegno che personalmente e come Gruppo sento di poter prendere, ma nello stesso tempo con un caloroso invito a non mortificare le regole che democraticamente ci siamo dati, perché chi rivendica costantemente il riferimento alla Costituzione deve anche capire ciò che da quella fonte primaria discende, ma in un modo non strumentale, bensì in un modo solo funzionale all'efficacia di un lavoro che è per la democrazia, per il Paese e soprattutto per chi, in questo momento, sta patendo più di tutti la crisi che stiamo vivendo.

il Movimento 5 Stelle solleva questione pregiudiziale e all'uopo propone di deliberare, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'atto Senato n. 941, in quanto il contenuto normativo del provvedimento in esame appare in aperto contrasto col dettato costituzionale riferito agli articoli 2, in quanto il contenuto normativo del provvedimento in esame appare in aperto contrasto col dettato costituzionale riferito agli articoli 2, 3, 9, 24, 32 e 41, consentendo il perdurante esercizio dell'iniziativa economica privata con modalità tali da recare danno alla sicurezza ed alla dignità umana, annientando la tutela del diritto fondamentale alla salute e all'ambiente salubre. Inoltre, la normativa in esame contrasta con gli articoli 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che proteggono il diritto di ciascuno all'integrità fisica e psichica ed alla salute. Vi è, inoltre, conflitto con il disposto dell'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il principio di precauzione, disatteso nella specie attraverso la legittimazione di attività comprovatamente dannose. Signori, voi tutti saprete che la sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2013 ha ha assicurato che un impianto industriale come l'Ilva può essere sì commissariato secondo il decreto-legge n. 207 del

fare ciò proprio in virtù dell'articolo 41. Ossia: «l'iniziativa economica privata è libera. Non può però svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge» - dice l'articolo 41 della Costituzione - «determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali». Quindi, la Corte costituzionale si è espressa nel senso dell'equilibrio tra l'attività economica e l'utilità sociale,

che sia indispensabile ed oggettiva la sussistenza di certe attenzioni da parte dell'impresa. Quindi, stiamo parlando di un'impresa che sta facendo, in modo reiterato, un danno all'ambiente, ossia di un'impresa palesemente fuorilegge.

facendo venir meno l'equo contemperamento di interessi, anche se nei decreti-legge predisposti per l'Ilva essi sono continuamente ed astrattamente enunciati. Ne risulta quindi privilegiata la produzione, seppur condizionata al rispetto e all'attuazione delle prescrizioni dell'AIA, ma in contrasto (quindi, in subordine) viene messa la salute che pure è un argomento tutelato dalla Costituzione (ce lo ricordiamo questo, no?). Inoltre,

oltre a sovrapporsi con altri articoli che tendono continuamente a deresponsabilizzare, si pone anche in contrapposizione

situazione, può anche essere chiusa. Per le fabbriche non commissariate questo vale, per quelle commissariate non vale più; basta mettere in atto un procedimento. Lo trovo gravissimo.

Questo garante che aveva funzioni di monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni dell'AIA e che doveva segnalare eventuali criticità ed idonee misure, una figura

e i criteri di liceità e di incompatibilità del commissario e del subcommissario e poi, con un ordine del giorno, presentato in ultimo dai relatori, addirittura di tutti

che questo signore è stato destinatario di una diffida ministeriale per mancata attuazione delle prescrizioni dell'AIA e della

volta a richiedere il parere del CNEL, ai sensi dell'articolo 98 del Regolamento. Ne ha facoltà. Il decreto-legge n. 61 disciplina, in via generale e con specifico riguardo allo stabilimento Ilva di Taranto, il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti per l'ambiente e per la salute, a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. decreto-legge è il terzo provvedimento d'urgenza adottato nel corso degli ultimi undici mesi per fronteggiare l'emergenza ambientale ed occupazionale dello stabilimento Ilva (forse tre sono un po' troppi). Esso fa seguito ai decreti-legge n. 129 e n. 207 del 2012. Emerge, dunque, in modo manifesto una violazione dei requisiti necessari per l'utilizzo della normativa d'urgenza da parte del Governo. La straordinarietà degli eventi, che solo giustifica l'utilizzo del decreto-legge, viene meno se si considera il fatto che il Governo nel breve periodo è dovuto intervenire più volte nell'ambito della stessa problematica. È necessario, inoltre considerare come per giunta è ragionevolmente ipotizzabile che anche le disposizioni previste dal presente decreto-legge non siano atte a risolvere definitivamente la questione in oggetto. È come se il Governo, in violazione dei requisiti di cui *ex* articolo 77 della Costituzione adottasse con decreto-legge alcune misure conscio della loro inefficacia, ne esaminasse in prima battuta gli effetti e le ripercussioni, ne riscontrasse le inefficienze a livello di applicabilità, le resistenze da parte delle forze politiche per poi reintervenire nuovamente, operando proprio sulle disposizioni più controverse o problematiche. Si tratta quindi di un sistema che permette, così, al Governo di correggere continuamente la rotta del proprio intervento legislativo, fino a soluzioni di equilibrio o di efficacia soddisfacenti. Un modello del tutto opposto rispetto a quello attuato dal legislatore ordinario che predetermina lo scopo da perseguire per mezzo dell'attività legislativa e che valuta, in via preventiva e non successiva (magari avvalendosi della fattiva collaborazione di tecnici), la compatibilità fra gli obbiettivi che si è proposto e gli effetti pratici che verranno a prodursi dall'entrata in vigore delle relative disposizioni; si segnala quindi come tale decreto-legge sia manifestamente incostituzionale perché viola il principio della libertà di iniziativa economica privata, riconosciuto dall'articolo 41 della Costituzione. La previsione di una procedura straordinaria di commissariamento, infatti, in assenza degli ordinari presupposti che la giustificano e, soprattutto, a prescindere dall'iniziativa dei titolari

in conclusione la disposizione di cui all'articolo 2-*ter*, inserita con proposta emendativa in sede di esame del presente disegno di legge di conversione del decreto-legge

viola il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto l'applicazione di tali norme pur se giustificata da motivazioni pratiche finalizzate al superamento della problematica in esame, crea, nei fatti, una palese disuguaglianza fra i cittadini residenti nelle altre regioni alle quali viene negata la possibilità di utilizzo di risorse proprie ai fini del rilancio della propria economia, della tutela dell'ambiente e della salute, del contrasto alla disoccupazione e del varo di misure atte a garantire un'adeguata efficiente od efficace predisposizione di iniziative delibera di non procedere all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 61, in materia di tutela dell'ambiente, salute e lavoro per imprese di interesse strategico nazionale. perché il caso creerà dei brutti precedenti, signora Presidente. Infatti, si dà priorità ad una situazione che, seppur gravissima, non è molto diversa da quanto accade in altre zone d'Italia: 39 siti di interesse nazionale e 18 di interesse regionale;

Tanti di questi, soprattutto al Nord, sono finiti nel totale disinteresse del Governo e dei *media*, siti per i quali non si propone lo sblocco del patto di stabilità regionale o locale e che producono forse gli stessi danni all'ambiente ed alla salute dei cittadini che vivono nelle vicinanze.

che ha creato disastri economici sia durante la gestione statale sia nel periodo di privatizzazione, e qui ricordo un nome e cognome, anzi, una sigla: IRI.

rottamatore di Firenze è stato anche proposto come candidato a Presidente della Repubblica! Stiamo attenti quindi, cari colleghi, a non creare situazioni già viste e che non fanno il bene dell'Italia.

Grazie, signora Presidente, grazie per l'attenzione, onorevoli colleghi. «la chiusura dell'altoforno e della cokeria delle acciaierie è una questione urgente. Sul piano dei danni ambientali, dell'inquinamento e della salute dei cittadini siamo già in ritardo»: non si tratta di parole incoscienti dette dagli ambientalisti di Taranto, né tanto meno dal Movimento 5 Stelle. A pronunciare queste parole fu, nel ruolo di direttore generale del Ministero, l'ex ministro dell'ambiente Corrado Clini ben dodici anni fa, in merito agli impianti dell'Ilva di Cornigliano a Genova. Su questa strada si è mossa la politica, verso impianti che producevano acciaio, verso impianti che per grandezza e capacità produttiva erano decisamente molto più piccoli dell'acciaieria di Taranto. A Taranto, invece, come ha risposto la politica in tutti questi anni? Colleghi senatori, siate onesti intellettualmente verso la città di Taranto, questo Stato si è comportato e continua a comportarsi in maniera vergognosa, non considerando la salute ed il futuro di una cittadinanza intera, tanto da esser sostituito più volte nel ruolo di ente che tutela i diritti dei cittadini e dei lavoratori da parte della magistratura. Il popolo tarantino ha udito dichiarazioni pubbliche sull'imminente ambientalizzazione dell'Ilva; affermazioni in cui si nega l'inquinamento della città e, se caso mai ci fosse, esso non è attribuibile ad industrie. I cittadini tarantini hanno visto videolettere postate su Internet in cui si affermava che l'inquinamento era sotto controllo e che la sfida per l'ecocompatibilità era vinta. Il tutto con politica locale e nazionale sostenuta da relazioni di pseudotecnici, tenuti sul libro paga dell'azienda. *(Brusìo).* PRESIDENTE. Aspetti un attimo, senatore, poi le ridarò anche dei minuti. Chiedo, per favore, un po' più di silenzio in Aula. Grazie. Abbiamo udito anche parlare di vocazione industriale di Taranto, senza neanche sapere quanto, con quella vocazione indotta da uno Stato incosciente e in seguito forzata da privati senza scrupoli, si violentavano e si ammazzavano le reali vocazioni di un territorio dalla storia plurimillenaria, baciato dal sole dorato e bagnato da un mare cristallino. Da ultimo, onorevoli colleghi, abbiamo udito il supercommissario arrivato in Commissione con l'intento di farci credere che Taranto è una sorta di Silicon Valley questo non vogliamo credere! Noi vogliamo dire che Taranto deve essere considerata il principale fallimento della politica italiana, perché siamo di fronte ad una realtà nella quale tutti hanno perso: ha perso la proprietà latitante o arrestata, i cui beni sono stati in parte sequestrati, beni che non si vogliono restituire alla comunità; hanno perso i lavoratori e i cittadini, miseramente posti in contrapposizione tra loro per una drammatica guerra tra simili; ha perso poi la politica, perché non ha saputo minimamente governare questa situazione; tutti hanno perso, tutti abbiamo perso! Ecco allora che noi abbiamo davanti la possibilità di riuscire a mettere a frutto il nostro impegno di politici e di cittadini solo se riusciremo a far convivere nello stesso tempo realtà produttive e comunità locali. Questa è l'unica sfida che abbiamo davanti, una sfida che al momento ci vede sconfitti; ma questa sfida non è un esercizio politico, non è pura teoria sociale, ma è la triste realtà. Avevate proposto in Commissione, con un emendamento, di iniziare il monitoraggio degli inquinanti nella zona di Taranto. Ma come iniziare? I dati ci sono: chiedete ai medici per l'ambiente, ad esempio; chiedete a chi la realtà la conosce, a chi quella realtà Come la vivono ad esempio Alessia, Federica, Pietro, Roberto e tanti altri bambini di Taranto, che hanno scritto parole che abbiamo il dovere di ascoltare, che voi, onorevoli senatori, avete il dovere di ascoltare e non

«Caro padrone dell'Ilva, vorrei che le fabbriche non inquinassero molto, perché questo provoca tante malattie e sofferenze. Anche i bambini che sono allergici, respirando tutto quel fumo delle fabbriche, stanno male. Caro padrone, pensa alla città di Taranto e al futuro di tutti noi. Costruiamo oggi un mondo migliore pieno di verde e senza inquinamento». Federica: «Vorremmo gridare tutti insieme al mondo intero che il veleno della città ci uccide e che desideriamo una città dove si respira vita, non morte. Grazie, Federica». «Ho nove anni» - dice Roberto - «e abito nel quartiere Tamburi di Taranto. Presidente, io ti invito nella mia città perché voglio che tu ci aiuti a combattere contro l'inquinamento e anche a costruire dove possiamo giocare». Dice Pietro: «È questo quello che vogliamo? Il fumo che inquina l'ambiente e la spazzatura che ogni giorno sporca sempre di più Taranto? O è questo quello che vogliamo: una città pulita e non inquinata? In questo modo possiamo aiutare l'economia di Taranto». Hanno poi detto i bambini della 5a D dell'istituto Rodari: «Le scriviamo perché speriamo che lei sia uno di quei pochi adulti che ascoltano i bambini. Siamo molto preoccupati per la nostra salute perché abbiamo letto sui giornali che ci sono tarantini di otto anni che hanno polmoni malati come persone di settanta anni che hanno fumato tre pacchetti di sigarette al giorno da quando erano ragazzini». *(Applausi dal Gruppo* «Fra di noi ci sono compagni che soffrono di allergia, asma ed altri problemi respiratori. Il nostro mare è considerato uno dei più belli d'Italia, ma non tutti sanno che per fare i bagni in estate siamo costretti a percorrere tanti chilometri nel traffico per raggiungere una spiaggia, dove l'acqua è sporca a causa delle numerose ville costruite a pochi metri dal mare che vi scaricano rifiuti. Il cielo di Taranto di notte non è splendente, perché i fumi delle nostre fabbriche lo ricoprono con tanto fumo grigio che nasconde le stelle. I nostri nonni ci raccontano di quando andavano al mare a piedi e facevano i bagni nel mar Piccolo e dei cieli stellati della loro infanzia. Noi facciamo fatica perfino ad immaginarli. Sappiamo che uno dei maggiori responsabili dell'inquinamento di Taranto è l'Ilva. Noi non desideriamo che la fabbrica chiuda perché molti nostri papà ci lavorano per mantenere le loro famiglie. Le chiediamo però: cosa dobbiamo scegliere tra salute e lavoro? Non sono tutti e due diritti garantiti dalla nostra Costituzione? Perché le fabbriche non possono utilizzare impianti di depurazione per offrire lavoro e salute? Vorremmo mangiare le nostre cozze crude, ma senza correre il rischio di ammalarci, come facevano i nostri nonni. Siamo sicuri che lei ci risponderà e perciò le chiediamo anche di dotare la nostra scuola di contenitori interni per consentire la raccolta differenziata dei rifiuti e di cassonetti esterni per poterli svuotare. Vedrà quanta carta un'intera scuola consumerà in un anno scolastico». Bene, da queste parole possiamo dire che sembra davvero che ci sia qualcuno che ha le idee molto più chiare di noi. Concludo allora il mio intervento con grande orgoglio di portavoce - forse per la prima volta da quando è iniziata questa avventura - per trovare oggi il coraggio di usare le parole giuste nel momento giusto. Noi del Movimento 5 Stelle al Governo un impegno affinché si adoperi per circoscrivere in modo più efficace e descrivere appunto con parole adeguate lo stato di calamità naturale di origine antropica, proprio a sottolineare tutti quei disastri ambientali che sono determinati dall'azione dell'uomo calamità naturali derivate da attività umane. È importante che questa tipologia di condizione ambientale venga oltremodo specificata, proprio per dare evidenza sociale di tutti quei fenomeni fortemente perturbativi, imputabili alla sola azione umana oppure ad un'azione congiunta di un fenomeno naturale ed un'azione umana.

fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, se dal fatto deriva la morte di più persone. quanto di propria competenza, l'esame delle iniziative recanti l'introduzione nel codice penale di un titolo espressamente concernente i delitti ambientali, con particolare riferimento alla previsione di specifiche fattispecie di «danno ambientale»,

mi hanno riportato a qualche anno fa, quando cercavamo in tutti i modi di far capire che la dialettica politica era importante, così come lo era rispettare la diversità di idee all'interno del Parlamento. Allora, invece, qualcuno la pensava diversamente e cercava di delegittimare coloro i quali la pensavano diversamente e cercava addirittura di ridicolizzare. Ma oggi, sentendo le parole del senatore Zanda, capogruppo del Partito Democratico, che stimo ed apprezzo, debbo dire che quella fase poco felice è tramontata e che la politica ritorna ad essere la politica con la p maiuscola. Un'altra riflessione ad alta voce la voglio fare nei confronti dei colleghi del Movimento 5 Stelle: persone perbene, che lavorano seriamente e concretamente. Qualcuno, però - ma dico qualcuno: proprio uno o due -, non è riuscito a fare il passo per diventare cittadino pubblico ed è rimasto cittadino privato. Questo mi amareggia.

a volte le emergenze trasformano in lusso qualche diritto fondamentale, almeno per un segmento di tempo sulla lunghezza della quale noi parlamentari dobbiamo vigilare affinché si possa ripristinare quanto prima quel diritto. Non possiamo stare a lungo in trincea, come «d'autunno sugli alberi le foglie», avrebbe detto il poeta Giuseppe Ungaretti nel 1918, scrivendo la poesia «Soldati». Per il disegno di legge di cui stiamo discutendo oggi dovremmo tener conto in modo esplicito degli articoli 4, 9 e 41 della nostra Costituzione e precisamente di alcune aporie emergenti dal confronto fra loro e di esse con lo sviluppo della conoscenza scientifica e tecnologica. La dialettica fra diritto al lavoro (articolo 4 della Costituzione) e libertà della iniziativa economica privata, purché non rechi danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (articolo 41), è una delle strutture invarianti, una costante, che caratterizza le società liberali moderne. Tuttavia, lentamente, ma in modo continuo e parallelo, nelle società aperte, si è sviluppata, emersa e distesa, una forza produttiva potente ed ora dominante. La scienza e le sue declinazioni tecnologiche hanno invaso e pervaso il panorama sociale. Il sapere scientifico è divenuto un'altra struttura invariante con la quale le società liberali dovranno articolarsi se si vogliono garantire i valori di dignità e benessere, libertà, uguaglianza e solidarietà. In questo scenario in cui la ricerca scientifica e tecnologica è una enorme forza produttiva che tende a dominare le altre (il lavoro, il capitale, le materie prime e le risorse energetiche), l'articolo 9 della nostra Costituzione (La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione) ci impone una sfida concettuale e politica. Tutelare il paesaggio ed il patrimonio della Nazione potrebbe costringerci a frenare lo sviluppo tecnologico; tutelare posti di lavoro e la libertà di impresa si scontra con la tutela della salute e con l'interesse strategico nazionale. Ecco che i tre articoli costituzionali, a cui il Governo coerentemente si appella nella prima riga del disegno di legge, diventano contrarietà interna e fra loro. L'emergenza ambientale, sanitaria ed occupazionale a Taranto e Statte è antica. Il contrasto fra difesa dei posti di lavoro e la salute degli stessi lavoratori,

Dov'è l'obbligatorietà dell'azione penale? Dove la responsabilità del magistrato accidioso? Ugualmente antico è il conflitto fra tutela ambientale e modello di sviluppo; era noto fin dagli anni Settanta quello della Montedison-Pertusola di Crotone, altrettanto quello delle acciaierie di Piombino, come dei siti industriali di Augusta e Marghera ancora più drammaticamente ed emblematicamente, a Seveso. Solo per citarne alcune fra le più note; note proprio perché furono e sono emergenze. emergenze. In genere, durante la prima Repubblica, quando un'azienda produttiva diventava di interesse strategico nazionale, i legislatori di allora mettevano in secondo piano i contrasti fra diritto al lavoro, tutela della salute e del territorio ambientale; a seconda degli interessi materiali in gioco e di impropri connubi oppure decidevano con procedure politicamente monche, lasciandoci in eredità appunto, terribili emergenze. Oggi, in questo secondo decennio del terzo millennio, non possiamo più permetterci il lusso delle mosse del cavallo nel gioco degli scacchi, scartando i problemi, spostandoci di lato per andare avanti. Per stare nella metafora, forse ci servirebbero le mosse perseveranti dei pedoni che coraggiosamente affrontano pezzi pesanti e trasversali come torri e re, obliqui e subdoli come gli alfieri ed i cavalli stessi. In uno scenario di elevata e crescente sensibilità e responsabilità civile (a volte anticipatrice di quella politica), abbiamo il dovere di ripensare il rapporto fra scienza, tecnologie e società; il nostro mestiere di parlamentari si dovrebbe distinguere proprio per tale *habitus* mentale:

salute, lavoro e acciaio, proprio come a Taranto. Un antico calabrese, che vorrei citare visto che sono stato eletto in Calabria, il pitagorico Assiopisto di Locri, attribuisce ad un mio altrettanto antico conterraneo, che cito perché sono di origine siciliana, Epicarmo di Iblea

e che, come disse un nostro connazionale, «tale» San Francesco d'Assisi: «Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile». Inventariare e monitorare le altre Ilva italiane per evitare di commissariale; istituire una commissione di inchiesta per mappare ogni sito produttivo di interesse strategico nazionale dove scienza e coscienza rischiano di rendere conflittuali e contrastanti gli articoli quattro, della nostra Costituzione, questo è un compito di ogni parlamentare e del Governo. Nell'attuale situazione di perigliosa concorrenza internazionale e di dominio della società meccanicistica e cartesiana, per rilanciare un settore economico sarebbe opportuno promuovere

questo è il mio auspicio per fare l'impossibile. **Testo Signora Presidente, ascoltando gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto viene da pensare che siamo sulla strada giusta. Da una parte, infatti, attraverso le espressioni che ha usato il Movimento 5 Stelle pensiamo di caricare sin fin da subito tutti tutti gli oneri, anche quelli non ancora dimostrati, in capo ad un'impresa che evidentemente altrimenti rischia di morire e non resterebbero che lo Stato e la comunità italiana a pagare i danni fin qui prodotti.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». Questo medesimo straordinario articolo dei nostri Padri costituenti che: «La legge» - (in questo momento siamo noi la legge, perché siamo i legislatori - «determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali». Credo che sia esattamente quello che stiamo

dilazioni all'indifferibile risanamento ambientale, per convincere Taranto, l'Italia, i mercati internazionali che la siderurgia può coesistere con il territorio circostante. Le migliori tecnologie applicate alle strutture d'impresa e il costante monitoraggio ambientale riusciranno a far convivere la produzione siderurgica senza che si creino ripercussioni sanitarie e ambientali, così come avviene peraltro in molte realtà europee (il caso Duisburg su tutti), divenendo fattore di buona occupazione, rispetto per i lavoratori, i cittadini e le imprese di quel territorio, oggi davvero martoriato da malattie, lutti, inquinamento e timori. Non compete però a noi emettere sentenze; a noi compete, come già stiamo facendo, ristabilire le migliori condizioni per aiutare la crescita e la competitività di questo e di altri settori produttivi. L'acciaio, come la chimica, il vetro e il cemento sono elementi essenziali per la catena industriale italiana e, se saremo capaci di ristrutturare come in questo caso, renderanno anche più verde l'economia italiana. L'obiettivo della *green economy* si ottiene attraverso un'adeguata revisione dei processi industriali, rendendoli rispettosi dei lavoratori e della realtà circostante; nel caso dell'acciaio anche attraverso un riciclo che vale il 100 per cento della materia prima, in considerazione del fatto che questo è il materiale più diffuso alla base del catena del valore di un prodotto. verso la produzione, però conformata alle *Best Avalable Technology* (BAT), cioè alle migliori tecnologie innovative e alle migliori pratiche industriali, è compatibile con le garanzie indispensabili per la salute e la qualità di un territorio sia urbano che agricolo. Potremmo sintetizzare affermando che non esiste possibilità reale di procedere alla messa in sicurezza degli impianti e alla bonifica del territorio interno ed esterno del perimetro dell'Ilva senza che l'Ilva mantenga la sua quota di mercato, orientativamente attorno agli 8 milioni di tonnellate,

I commissari Bondi e Ronchi, coadiuvati da una terna di esperti tecnici responsabili, sono coloro che dovranno comunicare a questo Parlamento, ogni sei mesi, come si muove la situazione di ammodernamento e di miglioramento della situazione esistente. Dunque ogni ipotesi diversa da questa consegnerebbe al Paese non solo un crollo dell'occupazione, che non saremmo probabilmente in grado di gestire in questo frangente di grave difficoltà economica e sociale, ma lascerebbe a debito pubblico oneri ambientali e sanitari spaventosi, che probabilmente non saremmo in grado di sanare di qui al prossimo futuro. la scommessa, quella che facciamo oggi insieme, è di trasformare un'impresa ad alto rischio sanitario ed ambientale in un soggetto virtuoso, promotore di occupazione, conciliando salute e ambiente. 2-*quater*, comma 3, si afferma infatti che i commissari, in accordo con la Regione e con gli enti locali interessati, promuovono iniziative di informazione e consultazione finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini, in conformità ai principi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale. A questo fattore di rispetto ed attenzione verso i cittadini, che diventa fattore culturale e di compartecipazione attiva al processo di miglioramento aziendale e ambientale in atto, si integra il rispetto delle disposizioni comunitarie, in conformità a quanto predisposto e richiesto dalla stessa Commissione europea nel 2012, a risoluzione delle procedure di infrazione già avviate presso la Corte di giustizia europea, predisponendo il piano aziendale che stiamo appunto autorizzando, che affronti e dia risposte per intero alle disposizioni AIA non ottemperate dalle imprese e la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento. Fondamentale in tal senso il ruolo di ISPRA ed ARPA, oggi investiti del ruolo di pubblici ufficiali garanti dei processi di modifica e risoluzione delle problematiche esistenti, nei tempi e negli obiettivi dati. È un passaggio storico questo, che induce tutti noi a riflettere su ciò che è stato reso possibile a causa dell'ignavia della politica e della speculazione economica. Ma - sia chiaro - non sarà questa un'autorizzazione a rimuovere responsabilità che rimangono intonse a carico dei soggetti imputati, pubblici e privati, coinvolti nella vicenda Ilva. Chi inquina paga e, con il presente disegno di legge, tutti i trattamenti economici e gli oneri di funzionamento della struttura commissariale sono per intero a carico dell'impresa. Una corretta, estesa e costante indagine epidemiologica, che contiamo venga attivata secondo il metodo SENTIERI, sarà poi conferma a posteriori che questo cammino di rinnovata serietà e correttezza aziendale, ma anche politico‑amministrativa, avrà prodotto

prima di sedere fra questi scranni ho sempre lavorato, in condizioni spesso anche disagiate, come semplice impiegata amministrativa. Spesso mi sono ritrovata a commentare la frase: «Non c'è mai fine al peggio». Mai però mi sarei sognata di lavorare qui come cittadina portavoce al Senato e mai mi sarei sognata che avrei pronunciato questa frase, proprio qui, proprio io in quest'Aula. E purtroppo non mi riferisco solo a questo decreto. Ebbene, sì, da quando è iniziato il nostro lavoro spesso ci siamo ritrovati a contrastare delle cosiddette prassi, che nulla hanno a che vedere con le modalità con cui un Parlamento dovrebbe legiferare e produrre atti per il bene del Paese. Spesso, anzi direi sempre, ci siamo ritrovati a lavorare e a discutere su provvedimenti del Governo che hanno solo l'intento di buttare fumo negli occhi, ma che in realtà non mirano minimamente alla soluzione dei problemi. Questo è quanto accaduto per la discussione di questo decreto-legge n. 61. Si parla di commissariamento: in pratica qualsiasi azienda di interesse nazionale (e ve ne sono molte come l'Ilva), che non ha rispettato le prescrizioni previste dall'AIA, che ha inquinato e sta inquinando, mettendo in pericolo la salute dei lavoratori e dei cittadini, e che rischia di essere chiusa, come sancisce il decreto legislativo n. 152 del 2006 (articolo 29-*decies*), può essere dichiarata commissariata. Quindi, in barba a tutte le normative vigenti, ha la possibilità, in base a questo provvedimento, di continuare a lavorare, sempre violando le prescrizioni dell'AIA, per altri 36 mesi. In questo modo si dà una via d'uscita a tutte quelle aziende che, pur violando la legge, vedono nel commissariamento la via di fuga. In pratica, questo decreto non è un salva Ilva ma è l'estensione del metodo Ilva a tutte le realtà industriali, e non per la tutela dell'ambiente, bensì per garantire la continuità produttiva delle stesse. Forse non ve ne rendete conto ma con questo decreto stiamo dando il via alla possibilità che quanto accaduto a Taranto si ripeta di nuovo, laddove sindaco, presidente della Provincia, Regione, Stato hanno regolarmente fatto le scelte sbagliate, con giri di parole, leggine regionali e accordi di programma che sono la dimostrazione dell'offesa all'intelligenza di un popolo intero. Il tutto con il favore di ignoranti politici locali e nazionali, sostenuti da relazioni di pseudotecnici tenuti sul libro paga dell'azienda che parlavano di vocazione industriale di Taranto senza neanche sapere, come ricordava il collega Lucidi, che stavano violentando e ammazzando le reali vocazioni di un territorio bellissimo come quello di Taranto. Sappiamo poi, invece, come sono andate le cose: sequestri degli impianti dell'area a caldo e perizie che affermavano che questo stabilimento produceva e produce eventi di malattia e morte. Nessuno dei suddetti signori si è ancora scusato con i padri, con le madri e con i figli di Taranto! Nessuno dei suddetti signori ha il coraggio oggi di mostrarsi pubblicamente a Taranto, così come nelle migliori abitudini dei peggiori vigliacchi!

e poi via, via, tutto l'*entourage* del partito unico e "tecnici" hanno perpetrato le violenze su Taranto a botte di decreti. Dapprima, a dicembre 2012, un provvedimento che di fatto ha salvato l'Ilva e ha condannato Taranto, stabilendo che in Italia la continuità produttiva è più importante della salute di cittadini e lavoratori. Stabilendo che un'autorizzazione integrata ambientale sarebbe stata sufficiente a tutelare la vita dei cittadini e degli operai, senza nessuna prova scientifica che potesse dimostrare che il problema degli eventi di malattia e morte si esaurisse. Stabilendo che l'illegalità in questo Paese non è solo un cattivo esempio ma una prassi consolidata, che permette alle aziende degli amici degli amici, nel momento in cui fossero accusate di non rispettare le leggi e la vita delle persone, di essere avvantaggiate rispetto a quelle che faticosamente, giorno dopo giorno, cercano di portare avanti la propria attività con onestà! Successivamente però la politica riesce a superarsi nella vergogna con un altro decreto - questo decreto - che stabilisce che la legge vigente sull'ambiente, che avrebbe portato ad una sospensione temporanea o totale dell'attività, è derogata! Che la famosa AIA - che la Corte Costituzionale ha accettato sulla fiducia come equilibrio tra il diritto al lavoro e il diritto alla salute, solo se fosse inderogabilmente rispettata - si potesse modificare e non certo in maniera più restrittiva. Un decreto in cui si nomina come commissario da parte dello Stato l'amministratore delegato dell'azienda privata che ora è commissariata e il quale commissario viene in anticipo sollevato da tutte le eventuali responsabilità! Ricordo che la valutazione di danno sanitario redatto dall'ARPA Puglia afferma che, semmai si rispettassero tutti le prescrizioni dell'AIA, il rischio di contrarre patologie non si annullerebbe, ma si dimezzerebbe solamente! Una vera tragedia per la salute dei cittadini, per i lavoratori e per i loro figli! Ma non solo, il Governo ha poca memoria e dimentica, nonostante la cittadinanza glielo ricordi continuamente, che le prescrizioni non rispettate dell'AIA, già certificate dall'lSPRA nelle due ispezioni fin qui effettuate, avrebbero dovuto essere sanzionate e che queste sanzioni, nonostante fossero decine e decine e reiterate in alcuni casi, non vengono ancora e a tutt'oggi imposte dallo Stato. Non sia mai che il privato si possa offendere? Eppure il M5S ha tentato tramite gli emendamenti di rendere il testo di questo decreto migliore, di proporre alternative: alternative frutto del lavoro portato avanti insieme con i cittadini di Taranto e non solo, con le associazioni, i comitati.

che le hanno stampate su una targa appesa in una via cittadina a ridosso dello stabilimento: "Nei giorni di vento nord-nord/ovest, veniamo sepolti da polveri di minerale e soffocati da esalazioni di gas provenienti dalla zona industriale Ilva.

ricordo a tutti che Taranto era la capitale della Magna Grecia e già nel IV secolo a.C. era considerata la più grande e la più ricca fra le città sul mare, prima obbligatoria tappa per chi dal mare Egeo si dirigeva verso Roma grazie alla sua felicissima posizione geografica. Una realtà come Taranto, complessa, ma anche dalle tante potenzialità, potrà rifondarsi solo a partire da una politica che faccia della partecipazione la regola da seguire, con rigore, nella quotidiana attività di Governo. La crisi di Taranto vive dentro la crisi italiana che, a sua volta, è parte di una crisi globale, ma Taranto non può vivere, oggi, senza acciaio, quando ogni altra alternativa economica (la cantieristica, lo sviluppo economico del porto, l'agricoltura, l'allevamento, la pesca, il turismo) segna il passo o comunque non decolla anche a causa dei processi inquinanti che hanno colpito la città e il suo territorio. Se il lavoro senza salute non è un diritto, è altrettanto vero che senza lavoro e senza mezzi di sussistenza non c'è dignità né c'è salute. Oggi è impensabile ricostruire il futuro, sperimentare un nuovo modello di produzione restando dentro lo stesso modello di sviluppo, incompatibile con la natura e dunque con la vita. L'età dell'acciaio - metallo prezioso che muoveva automobili, carri armati e frigoriferi, intelligenze e lavoro di milioni in tutto il mondo - non è però finita. I metalli, più o meno preziosi, non servono soltanto a costruire merce del passato, energivora e inquinante ma anche gli oggetti simbolo di un nuovo modello di sviluppo, come i pannelli solari, le pale eoliche, che hanno molto a che fare con la trasformazione industriale dei metalli e con la sostenibilità dello sviluppo energetico. La conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, è il quarto provvedimento, adottato nell' ultimo anno per fronteggiare l'emergenza ambientale ed occupazionale dello stabilimento Ilva di Taranto a testimonianza degli enormi sforzi compiuti a salvaguardia dell'occupazione, ma anche dell'ambiente e della salute

passata dei precedenti decreti e delle pronunce dell'autorità giudiziaria e della stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 85 del 2013. Oggi, il terzo decreto-legge, n. 61, cerca di effettuare un equo contemperamento tra i principi costituzionali relativi alla tutela del lavoro, alla alla salubrità dell'ambiente, alla salute pubblica, alla libertà dell'iniziativa economica ed alla tutela della proprietà. E per la prima volta viene affermata la connessione tra l'impiego delle somme sequestrate e il piano di recupero ambientale e il piano industriale, accogliendo il principio per la prima volta in Italia «di chi inquina paga», più volte richiamato dalla direttiva sulla responsabilità ambientale. E con il superamento della figura del garante ci sarà anche la giusta rivalutazione delle agenzie ambientali pubbliche, di livello regionale o nazionale, che risultano più funzionali alle finalità da conseguire. Il professor Assennato, direttore dell'ARPA, ha riferito in sede di audizione che la collaborazione tra le due agenzie è stata perfetta. Entrambe infatti attraverso controlli tipici di un sistema agenziale autonomo, non sottomesso quindi al potere politico o alla musica del Governo, come qualcuno ha ironicamente scritto per l'ARPA, garantiranno anche grazie alle attività ispettive dell'ISPRA, con la qualifica di polizia giudiziaria, quella necessaria autonomia che sarà o meglio garante della legge nei confronti della collettività. Tutto questo a conferma della capacità di questo Parlamento e di questo Governo di fare, ma anche di saper fare, scongiurando un evento traumatico quanto irreversibile come lo *stop* alla produzione e lo spegnimento degli impianti, che segnerebbe la fine non solo di un polo industriale e di una intera città, ma della siderurgia italiana, sia a Sud che al Nord, e, cosa ben più grave, la bonifica del territorio. Basti qui ricordare che l'impianto produce il 75-80 per cento del PIL di Taranto ed è il garante dell'autonomia In caso contrario, sarebbero lacrime amare per la nostra bilancia commerciale per una eventuale importazione da Paesi come India, Germania o Cina, che con la sua produzione copre il 50 per cento della produzione totale, contro il 20 per cento di quella europea, metà della quale si produce in Italia (9 per cento circa). Ci sono in gioco 11.431 posti di lavoro diretti, 3000 indiretti, altri 20.000 che dipendono dalle cokerie e dalla lunga filiera produttiva dell'Ilva. Ma ancora non basta, lontano da Taranto ci sono altri quattro stabilimenti italiani e un paio all'estero, privi di lavorazioni a caldo, che dipendono per il loro lavoro di trasformazione da questi altiforni. È difficile quantificare, ma c'è chi parla di 100.000 salari italiani legati direttamente o indirettamente al cammino E312 e al resto della

al lavoro e alla salute ha una storia lunga che inizia ben prima dell'Ilva di Taranto. Viene da lontano, dall'Italsider, dagli impianti chimici di Porto Marghera, dall'Acne di Cengio, da altri impianti inquinanti in Liguria, in Puglia, in Toscana, in Campania, e proprio in Campania la chiusura dello stabilimento doveva essere l'inizio della rinascita dell'aerea di Bagnoli, un gioiello del Mediterraneo, dopo i sigilli alla produzione siderurgica, ma a vent'anni di distanza ancora si aspetta il risanamento dell'aerea dai veleni industriali. L'unica strada per tentare di salvare lavoro, economia e salute è quella di liberarsi dal gioco di chi si è reso responsabile del disastro di Taranto, facendogli pagare i costi della bonifica. Nella terza settimana di maggio è stato effettuato questo sequestro di 1,2 miliardi di euro prima e di 8,1 miliardi dopo, frutto del risparmio sulla sicurezza dei lavoratori, sull'ammodernamento degli impianti e sulla salute di 200.000 cittadini. Un capitale enorme che, come hanno scritto i giornali, vale il doppio dell'intero gettito IMU e che, secondo gli stessi magistrati, dovrebbe essere utilizzato per un risanamento coatto dell'Ilva. Se il diritto al lavoro e alla salute fossero stai presi sul serio all'Ilva, e prima ancora all'Italsider, non ci saremmo trovati nell'attuale situazione disastrosa da un punto di vista sociale e ambientale. Voglio pertanto ribadire che solo la continuità produttiva potrà essere condizione essa stessa del risanamento ambientale. Mai come in questo caso è necessario ragionare non in termini contrapposizioni ideologiche ma piuttosto in termini di convergenza ideologica o, addirittura, di confluenza ideologica, la soluzione offerta dal provvedimento di una gestione commissariale straordinaria è ispirata alla medesima logica di una gestione intergrata tra le esigenze ambientali e quelle occupazionali. È il caso di Linz in Austria e più ancora di Duisburg in Germania, dove l'impianto della ThyssenKrupp ha una produzione raffrontabile a quella di Taranto, eppure gli interventi fatti in materia ambientale e di sicurezza la rendono perfettamente compatibile con la vicinissima città. I dati OCSE ci confortano nella strada intrapresa, la domanda mondiale d'acciaio dovrebbe aumentare a 2,3 miliardi di tonnellate entro il 2025, grazie principalmente alle costruzioni, ai trasporti e all'ingegneria meccanica, sopratutto nelle economie emergenti. È essenziale che l'industria siderurgica italiana possa concorrere approfittando di queste opportunità di mercato. La stessa Commissione europea ha predisposto un nuovo piano strategico per il settore siderurgico. L'Italia ha bisogno del settore siderurgico per aiutare la crescita e la competitività di altri settori produttivi. Settori come l'acciaio, la chimica, il vetro e il cemento sono elementi essenziali di una catena del valore industriale capace di rendere più verde l'economia. L'acciaio stesso è riciclabile al 100 per cento ed è il materiale più diffuso alla base della catena del valore di un prodotto. Cari colleghi,

...che sarà il più avanzato in Europa in termini di compatibilità ambientale. Non sarà la svolta a rischio zero, ma potrebbe avvicinarsi. Grazie a questo provvedimento possiamo avere anche noi l'orgoglio di avere contribuito, nella misura delle nostre forze, a tale cambiamento. Mi auguro che questo Governo, signor Sottosegretario,

il senatore è assente, ma mi preme raccontare un episodio che è avvenuto mentre ero in Commissione bilancio in attesa che arrivasse il nostro Presidente. Mi sono sentita dire da un onorevole collega: «Beh, tu e il tuo *leader* portate i 1.600 morti e i malati sul palco. Vai a conquistare gli elettori così». Era il senatore Guerrieri Paleotti

Grazie.

Prenderemo in considerazione ciò che è avvenuto. È iscritta a parlare la senatrice Gambaro. Ne ha facoltà. *(Il senatore

alla calma. Chiedo che l'Aula torni ad essere rispettosa di tutti - insisto - nel linguaggio e nei comportamenti fisici. *(Misto)*. Signora Presidente, i Governi che si susseguono adottano una particolare solerzia per i provvedimenti che garantiscono la sopravvivenza delle aziende e della produzione, mentre posticipano, se non omettono del tutto, le azioni a tutela della salute. Certo, le esigenze e le necessità di tipo industriale e occupazionale spingono chi deve amministrare e l'opinione pubblica verso soluzioni che abbiano come obiettivo prioritario quello della salvaguardia dei livelli di produzione e dei posti di lavoro. Chi direbbe che questa urgenza pubblica da soddisfare non è di primaria importanza? In dodici mesi, i due ultimi Governi (Monti e Letta) hanno varato due decreti salva Ilva e nominato un Garante per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui chiediamo il ripristino, visto che questa figura è stata soppressa nella versione del decreto approvata alla Camera, un commissario straordinario (Enrico Bondi, già amministratore delegato dell'azienda), un sub-commissario (Edo Ronchi) ed un comitato di tre esperti. tutto questo, eppure non sono riusciti ancora a bloccare le emissioni nocive che dallo stabilimento siderurgico si diffondono sul vicino quartiere Tamburi e sui territori dei Comuni di Taranto e Statte. Ho avuto modo la scorsa settimana di prendere parte alla delegazione parlamentare all'Ilva di Taranto. Ho visto i luoghi, esaminato dati epidemiologici attendibili e parlato con la gente del posto. Il problema sanitario è di enormi dimensioni e non può essere più disatteso dalle autorità competenti. I riscontri scientifici sull'incidenza degli agenti cancerogeni presenti nell'atmosfera di quella zona della Puglia e l'insorgenza di malattie legate alle emissioni dei fumi tossici sono davvero allarmanti. A questo punto non c'è più margine di errore. Ho ascoltato considerazioni tecniche e letto perizie e valutazioni ambientali molto discordanti rispetto all'asse centrale e alle prospettive concrete della norma in esame. L'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale, ovvero l'insieme delle prescrizioni stabilite dal Ministero dell'ambiente per abbattere l'inquinamento dell'area a caldo (parchi minerali, cokerie, altiforni e acciaierie), è il fronte più delicato per l'Ilva. D'altra parte, l'azienda è stata commissariata il 4 giugno dal Governo poiché sull'AIA è in netto ritardo sui tempi, così come hanno accertato nelle diverse ispezioni fatte dai tecnici dell'ISPRA. Sempre per l'AIA, l'Ilva annuncia che «sono state avviate misure per il contenimento immediato dell'impatto ambientale sia per le emissioni convogliate sia per quelle diffuse»; inoltre, «si è installata una rete di rilevamento e monitoraggio delle emissioni (ad esempio, rete di rilevazione, rete idranti dei parchi, sistemi di nebulizzazione) e sono stati emessi i primi ordini

come Bondi ha annunciato il 23 luglio scorso nell'audizione al Senato (dinanzi alle Commissioni riunite 10a e 13a), della revisione già intrapresa dall'azienda. Ad ogni modo, auspico che nel *mare magnum* dei provvedimenti emanati, delle battaglie senza soluzione di continuità tra le autorità amministrative e giudiziarie e tra gli enti competenti e le associazioni ambientaliste, che si sono sommati, incrociati e scontrati sulla vicenda, questo provvedimento sia dirimente e costituisca un punto di partenza utile a far fronte allo stato di necessità medico e ambientale perdurante ormai da anni. Richiediamo inoltre che venga ripristinata la valutazione sull'impatto sanitario. Essendo l'Ilva il centro di produzione siderurgica più importante d'Europa e proprio al centro degli snodi marittimi commerciali del Mediterraneo, l'impianto di Taranto ha assunto una rilevanza notevole anche da un punto di osservazione internazionale. Ricordiamo che le AIA rilasciate nel 2011 erano già in contrasto con la direttiva europea 2008/1/CE. Dobbiamo considerare che una risoluzione efficiente del caso Ilva non è dunque rilevante solo per il futuro dei polo siderurgico tarantino, ma anche nella valutazione dell'affidabilità estera dell'Italia, sia nella gestione delle procedure di autorizzazione e controlli ambientali delle imprese industriali, sia nella coerenza con le direttive ed i regolamenti dell'Unione europea.

Presidente, illustri colleghi, rappresentanti del Governo, onorevoli cittadini, la questione dell'Ilva di Taranto costituisce l'emblema di ciò che è stato il ruolo dello Stato, anche negli ultimi vent'anni, nella politica industriale del nostro Paese e, segnatamente, del Mezzogiorno d'Italia. La città di Taranto è stata per anni illusa dai nostri Governi di poter proseguire, in rinnovate forme privatistiche, un cammino di sviluppo economico solido e duraturo e si trova oggi invece a dover scegliere tra la salute dei propri bambini e la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali minimi di un'area peraltro già fortemente provata da una difficile crisi economica e sociale. le misure proposte dal Governo - peraltro imposte dalla complessità delle iniziative giudiziarie in corso - sono un'ulteriore pagina di una visione politica precaria e provvisoria, inidonea a ridisegnare un serio progetto di sviluppo e di rilancio del territorio interessato. Trova inequivocabile conferma l'aridità politica di questo Governo. Occorre invece iniziare a immaginare concretamente un futuro nuovo per l'intera area tarantina che, pur nel rispetto dei bisogni del mondo del lavoro, sappia incentrare il proprio impegno sulle risorse vere del territorio, come il mare, la cultura e il turismo. In questa prospettiva serve una visione politica coraggiosa e nuova. Il reddito di cittadinanza, che ieri in quest'Aula è stato respinto con pareri e voti contrari del Governo e dal PD con e senza "L", può rappresentare lo strumento innovativo idoneo ad assicurare maggiore serenità nell'affrontare una problematica in cui troppo spesso, sull'altare degli interessi della grande industria e di qualche politicante da strapazzo, si sono sacrificati i diritti fondamentali delle persone, fra cui primariamente la salute, specie L'invito, in altri termini, rivolto a tutte le forze politiche, di destra e di sinistra, è di non continuare ad affrontare il problema dell'Ilva di Taranto con la logica di chi ricerca un contingente consenso elettorale o, peggio, la benevolenza di qualche gruppo industriale. Sul punto è sufficiente ricordare le vergognose affermazioni di Bondi sull'inquinamento a Taranto per comprendere come, anche in questa ipotesi evidentemente, le categorie dell'avere continuino a suscitare un fascino spesso irresistibile, ovvero gli *slogan* elettorali dell'attuale Presidente della Regione Puglia, aspirante poeta, che recitavano: "Cambia l'aria tarantina con la legge antidiossina". *(Richiami Oggi più che mai, specie alla luce dei recentissimi dati sui gravissimi danni alla salute che hanno colpito in questi anni la cittadinanza dell'area tarantina interessata, la politica deve assumersi le proprie responsabilità e, *in primis*, quella di avere coraggio nel tracciare nuovi orizzonti di sviluppo economico e sociale, anche quando ciò possa comportare nell'immediato scelte impopolari. Anche per queste ragioni il presente decreto non costituisce e non può costituire la risposta giusta ai bisogni dei cittadini.

il provvedimento in esame rappresenta senza dubbio un tassello importante del complesso percorso di risanamento e di riadeguamento di una delle realtà economico-industriali maggiormente strategiche del nostro Paese. Voglio rinnovare pertanto la mia soddisfazione nei confronti di questo provvedimento e verso gli aspetti che in esso sono stati introdotti anche alla luce delle recenti letture parlamentari. Si tratta infatti di uno strumento indispensabile di intervento che si colloca in una delle pagine più complesse della storia industriale italiana. Il problema dell'Ilva, come sappiamo bene, non si limita a pochi aspetti e non si limita al solo impianto di Taranto. Le questioni che lo stesso Governo è stato chiamato ad affrontare sono molteplici. il piano di intervento, rappresentato da tre distinti decreti-legge che si sono avvicendati nell'ultimo anno, danno la dimensione di quanto la cognizione dell'urgenza e della volontà corale di intervento siano state indispensabili. Il provvedimento di oggi è dunque parte di un percorso che si è sviluppato in anni di confronto istituzionale, di polemiche e di esasperazioni sociali, ma che sembra orientarsi - finalmente - verso un processo di armonizzazione economico-ambientale, rappresentato dall'attuazione di un commissariamento, da considerarsi condizione indispensabile per l'emancipazione dell'impianto e per la sua stessa sopravvivenza. Il provvedimento infatti è volto proprio a disciplinare il commissariamento straordinario di uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, la cui attività produttiva comporta pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute, a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Il provvedimento opera degli importanti passi in avanti disponendo la delibera del commissariamento di tutti gli impianti siderurgici della società Ilva Spa, annoverandoli tra quelli di interesse strategico nazionale, a norma dell'articolo 1 decreto-legge n. 207 ed attribuendo al commissario e al subcommissario poteri per i piani e le azioni di bonifica previsti dall'AIA. Di conseguenza, al commissario viene anche riconosciuto un importante ruolo di confronto con le istituzioni e con le comunità locali. Un orientamento di pragmatismo e di lungimiranza che sicuramente si colloca in una fase nuova del processo di risanamento. Appare opportuno evidenziare che il provvedimento risulta innovativo anche perché, per la prima volta, si configura l'ipotesi di commissariamento di un'azienda per ragioni connesse al risanamento ambientale. Sebbene sia stata oggetto di numerose critiche la modalità con cui si è proceduto all'individuazione dello stesso commissario straordinario, che collima con la figura dell'amministratore delegato scelto dalla proprietà, le ragioni di opportunità, di celerità e di pragmatismo dovuti anche all'eccezionalità della fattispecie affrontata ci hanno imposto il superamento di ogni ulteriore reticenza. In questa prospettiva merita anche attenzione quanto introdotto nella lettura alla Camera del provvedimento stesso: infatti nella procedura del commissariamento ci deve essere l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, rinnovando un coinvolgimento attivo del Parlamento nelle dinamiche di intervento di risanamento di un'azienda altamente strategica per il nostro Paese. Un ruolo, quello del Parlamento, che deve considerarsi fondamentale e di riferimento, soprattutto se si tiene conto delle misure che si apprestano ad essere intraprese nella fase di commissariamento e che risultano articolate e particolarmente importanti per il futuro e le potenzialità dell'impianto siderurgico. Quanto evidenziato in sede di audizione dal commissario straordinario Enrico Bondi delinea tra l'altro i prossimi *step* operativi ai fini del risanamento degli impianti e, tra questi, la mobilitazione ed il rafforzamento delle risorse aziendali dedicate al risanamento: la verifica dello stato di attuazione dell'AIA, delle prescrizioni della magistratura e degli organi di controllo, ed il supporto della predisposizione e della realizzazione del nuovo piano di interventi ambientali, al fine di renderlo connesso ed integrabile con il piano industriale. Per questa ragione, ed avremo modo di chiederlo anche attraverso un ordine del giorno, sarebbe auspicabile consentire il monitoraggio delle attività connesse al commissariamento straordinario, considerata l'articolata e strategica natura delle stesse, attraverso la presentazione di una relazione sullo stato di attuazione delle misure previste dal provvedimento alle Commissioni parlamentari competenti da parte del commissario straordinario e del subcommissario, proprio per preservare questo rapporto di funzionalità operativa tra commissariamento, impianto e istituzioni, che - come abbiamo visto - ha rappresentato la strategia più adeguata per superare un'*impasse* che sembrava priva di soluzioni percorribili sul breve periodo. Ma sarà anche nostra cura rivolgere un'ulteriore riflessione al Governo proprio sul versante delle dinamiche e delle modalità di esecuzione delle bonifiche dell'impianto. È a tutti nota la complessità dei processi di bonifica di un impianto come quello di Taranto, soprattutto perché devono essere avviati mantenendo l'utilizzo produttivo del sito e allo stesso tempo garantire una certa celerità nelle stesse operazioni. Riteniamo sia indispensabile che ad operare in questo comparto siano aziende ove possibile italiane e non aziende estere, per quanto queste siano competenti e specializzate in questo delicato settore. Questo per garantire una sorta di coerenza con la *mission* che in fondo sottende l'intero programma di intervento di risanamento che mira a ricollocare il sistema produttivo italiano in una cornice nuova e proficua, evitando nel contempo che iniziative caratterizzate da alti livelli di coinvolgimento operativo con forti riflessi sulle potenzialità future dell'impianto e in generale dell'industria italiana siano paradossalmente vincolate ad interlocutori esteri. In questo senso si commetterebbe un grave errore. Ma il percorso di intervento sull'impianto di Taranto, sappiamo bene, è stato condizionato anche da molte ombre che hanno sistematicamente rallentato le dinamiche di risanamento. Ricordiamo il sequestro dell'area a freddo dello stabilimento e dei prodotti finiti da parte del gip di Taranto nel novembre 2012, un'iniziativa coincidente con la data prevista per l'avvio, da parte dell'Ilva, delle attività stabilite dal piano degli interventi della nuova AIA. Dunque un conseguente rallentamento del programma di risanamento ambientale che ha messo a rischio sia le misure per la protezione dell'ambiente e della salute, sia la stessa continuità produttiva. In questo scenario si è collocato il precedente intervento legislativo - convertito con la legge n. 231 del 2012 - che, recependo la nuova AIA, ha stabilito le misure sia per il monitoraggio delle iniziative della società finalizzate all'attuazione delle prescrizioni di AIA, sia le sanzioni pecuniarie ed amministrative in caso di inadempienza. Questa legge ha rappresentato senza dubbio l'inizio di questa fase nuova, consentendo l'avvio del piano degli interventi per il risanamento ambientale dello stabilimento, nonostante l'opposizione della procura e del gip presso la Corte costituzionale contro la legge stessa. Nell'aprile del 2013, la Consulta ha respinto le eccezioni di incostituzionalità sollevate dalla procura della Repubblica e dal gip di Taranto, rilevando peraltro che le misure di risanamento ambientale dello stabilimento corrispondono all'obiettivo della salvaguardia contestuale del diritto al lavoro e del diritto alla salute. Pertanto, il decreto-legge in esame rappresenta anche lo strumento attraverso il quale si è inteso dare continuità attuativa alla legge n. 231 del 2012 anche alla luce delle motivazioni della sentenza della Consulta. Non dimentichiamo che il decreto-legge ha un obiettivo ambizioso, quello di armonizzare più aspetti dello stesso problema: potenzialità economiche, diritto del lavoro, tutela ambientale e della salute. Elementi che possono sembrare confliggenti e le cui modalità di tutela non hanno visto sempre un consenso trasversale. Ma il provvedimento ha dimostrato che una rinnovata mentalità nelle dinamiche di intervento e di rettifica dell'operatività di un sito industriale o di una qualsivoglia realtà produttiva che presenta delle criticità può condurre a risultati proficui. Come è stato chiaramente evidenziato anche in occasione della discussione nelle Commissioni competenti, il decreto può tranquillamente configurarsi come una pratica di eccellenza potenzialmente applicabile in casi simili. Questo ultimo *step* del percorso di ripristino sostenibile dell'Ilva è una metafora della capacità di intervento del sistema Italia e di come questo possa essere riadeguato pregevolmente alle esigenze mutevoli del Paese. Tutto deve ruotare intorno ad una rinnovata mentalità ambientalista del Paese, che sappia superare i pregiudizi e soprattutto determinate costrizioni alimentate più da pressioni ideologiche - per arrivare ad una nuova stagione dove, come dicevo, la crescita economica non può confliggere con un reale sviluppo sostenibile dei processi produttivi. grazie.

attraverso il quale, oggi a Taranto e domani anche in altri stabilimenti, può essere garantita una sostanziale impunità ai commissari straordinari e agli incaricati da Più precisamente, leggendo il testo dell'articolo, si capisce che la mera predisposizione formale del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per il rispetto delle prescrizioni dell'AIA, di cui al comma 5, e del piano industriale di conformazione

illeciti» - leggo testualmente - «strettamente connessi all'attuazione dell'AIA e» - attenzione - «delle altre norme a tutela dell'ambiente e della salute». Quindi, non stiamo parlando solo del rispetto formale delle prescrizioni AIA, che sappiamo essere violate ancora oggi. I membri della Commissione ambiente del Senato che hanno visitato gli stabilimenti credo una settimana fa (o poco meno), hanno riscontrato con i loro occhi la presenza di discariche e di emissioni fuggitive, la assoluta inefficacia di sistemi di abbattimento del particolato di carbone quali questi dell'innaffiamento, che veramente sembrano essere totalmente inefficienti.

come Nazione, ai cittadini tarantini che ancora stanno pagando un prezzo carissimo (e non solo loro). *(Applausi

portati avanti dai colleghi quando si sta affrontando un provvedimento che riguarda l'Ilva di Taranto, il cui proprietario è il signor Riva, e fanno riferimento a fatti notori (non cito nessuno)... Riva è corretto.

ci dispiace molto che l'Aula sia abbastanza vuota durante questo dibattito, perché il provvedimento in esame è estremamente importante e - soprattutto - perché ci dovrebbe far confrontare davvero in modo approfondito su un tema che è quello dell'idea di sviluppo

noi abbiamo avuto, in anni e anni, un intervento che è stato assolutamente C'è stata una prevalenza, senza alcun tipo di limite, delle esigenze della produzione, di un'idea di uno sviluppo bacato, rispetto a quello che era il diritto alla salute dei cittadini,

in contrasto con il decreto precedente, che, a nostro avviso, non era in grado di affrontare le questioni drammatiche dell'Ilva e, quindi, dell'ambientalizzazione, della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini e dei lavoratori. Era un decreto a nostro avviso ancora una volta compiacente con la proprietà dei Riva. Come SEL abbiamo voluto questo decreto perché pensavamo - e pensiamo - che il commissariamento fosse

Per la prima volta avevamo l'occasione di concretizzare e mettere alla prova l'articolo 41 della nostra Costituzione. Invece riteniamo che sia stata un'occasione persa perché, ancora una volta, non si è avuto il coraggio di coraggio di avere in mente solo e unicamente l'interesse pubblico e l'interesse di Taranto, ed è stata introdotta una serie di

non solo siano attuate le prescrizioni dell'AIA, ma soprattutto che si assicuri nel modo più compiuto possibile la sostenibilità la sostenibilità ambientale e sanitaria della produzione, obbliga, se davvero si vuole fare questo, a mettere in campo innovazione tecnologica, la capacità anche di mettere in campo un *know-how* che sarebbe fondamentale ai fini dell'ammodernamento dell'ammodernamento dei sistemi di produzione dell'acciaio e che forse, se l'impresa fosse stata più lungimirante, avrebbe potuto renderci più competitivi in Europa e nel resto del mondo.

chiedo come si fa - lo dico qui con chiarezza, l'ho detto in Commissione, abbiamo provato a far ragionare - a non comprendere che vi è un'incompatibilità oggettiva.

proprio perché si è scelto di nominare commissario straordinario Bondi. Quindi, da una parte abbiamo l'incompatibilità e dall'altra ci troviamo di fronte all'eliminazione di una figura che era il garante per l'attuazione dell'AIA,

trovo anche grave che nell'ordine del giorno che la maggioranza ha approvato, dopo aver di fatto deciso di ritirare i suoi emendamenti e di dichiarare inemendabile il decreto-legge in Commissione, in Commissione, essa non si sia neanche fatta carico della possibilità di prendere in esame in un successivo provvedimento il fatto di poter reintervenire sulla questione del garante.

questo lo trovo grave, perché nel momento in cui ci sono legislazioni avanzate da questo punto di vista (quindi non c'è più soltanto l'AIA, non c'è più soltanto la valutazione d'impatto ambientale, ma anche la valutazione d'impatto d'impatto sanitario), con un emendamento del Governo - gravissimo - si fa in modo che questo sia inefficace e non se ne debba tener conto, stabilendo una metodologia (quella di un decreto-legge) che non è certamente quella riconosciuta anche a livello europeo.

oppure fare in modo che le sue prescrizioni non siano attuate completamente. L'AIA deve essere implementata, migliorata, si può renderla più efficace e questo deve essere il compito

ai cittadini e ai lavoratori, e immediatamente si fa in modo che questa occasione sia perduta. Io vi invito ancora una volta; avete ancora l'occasione per poterci ripensare e per fare in modo che davvero questo primo commissariamento sia un segno di svolta, non solo per l'Ilva, ma per tante altre fabbriche che stanno attendendo. Riguardatevi la graduatoria che è uscita qualche giorno fa sull'incidenza dei tumori: Taranto, Porto Marghera, Civitavecchia. Riflettiamo, è ora di dare una spinta, perché rispettare l'ambiente e la salute dei cittadini e dei lavoratori significa anche fare una grande operazione di innovazione tecnologica. Questo è lo sviluppo che vogliamo.

colleghi senatori, il Governo è intervenuto con il decreto‑legge n. 61 del 2013 per far fronte ad una situazione di emergenza conseguente al sequestro preventivo dei beni di proprietà dei signori Riva; un sequestro, come tutti sappiamo, che ha un valore di 8,1 miliardi di euro. È una situazione questa, signor Presidente, che rischia di provocare la chiusura degli stabilimenti dell'Ilva, e non solamente dell'Ilva di Taranto, ma anche delle aziende collegate su tutto il territorio nazionale. La società Ilva tiene a Taranto tutte le lavorazioni a caldo, che sono quelle maggiormente inquinanti di tutta la filiera Si tratta di un'iniziativa industriale altamente impattante per il territorio, che per quarant'anni ha continuato ad inquinare il suolo, le falde idriche e la qualità dell'aria, senza che venissero prese adeguate misure di sicurezza per l'ambiente e per la salute pubblica. Se è vero che una maggiore sensibilità verso le tematiche ambientali è nata solo negli anni Novanta, è altrettanto vero che negli ultimi decenni la società Ilva non ha fatto niente - e ripeto: niente - per adeguare l'impianto alle migliori tecniche disponibili e all'autorizzazione AIA. Tuttavia, nonostante i persistenti interventi della magistratura, che solo negli ultimi due anni sembra essersi ricordata delle criticità ambientali di Taranto e del quartiere Tamburi, tutti concordano sulla necessità di proseguire l'attività industriale dello stabilimento di Taranto, sia per motivi occupazionali, sia per poter assicurare l'effettiva realizzazione degli investimenti occorrenti per il risanamento ambientale dell'area ed evitare il ripetersi di una situazione simile a quella di Bagnoli. Ho ricordato al presidente Vendola, nell'incontro che ha avuto luogo in prefettura quando siamo andati in missione con le due Commissioni competenti, il fatto che l'Ilva di Taranto si vede dal satellite molto meglio che la Grande muraglia in Cina. Pertanto la situazione dell'Ilva è particolare, sia per la struttura aziendale e i connessi risvolti occupazionali diffusi su tutto il territorio nazionale, sia per la criticità ambientale dell'area e per l'estensione territoriale dell'inquinamento, ed è unica nell'ambito del settore siderurgico italiano. Questa è la cronaca. In dodici mesi due Governi, Monti e Letta, sono stati capaci di varare tre decreti «salva-Ilva», di nominare un garante, di nominare un commissario straordinario, di nominare un subcommissario, un comitato di tre esperti e una squadra infinita di consulenti, ingegneri e tecnici. un anno speso in battaglie istituzionali e giudiziarie, un anno di conflitti tra periti, giudici e ambientalisti; un anno in cui nulla è cambiato, signor Presidente, o quasi nulla è cambiato. Un anno che è servito solo ad aumentare la rassegnazione e la paura tra la popolazione tarantina. Come Gruppo Lega Nord, siamo stati molto critici nei confronti di tutti i provvedimenti "ad aziendam" emanati per l'Ilva, l'Ilva, perché riteniamo che il commissariamento sia da limitare solo allo stabilimento di Taranto ‑ e, per l'amor del Cielo, teniamo lontano da questa vicenda il signor Prodi; la prego, signor Presidente, si faccia carico di questa cosa ‑ e perché abbiamo chiesto al Governo di estendere lo stesso provvedimento anche agli altri siti presenti al Nord. Ci sono molti emendamenti, presentati anche al primo decreto, che prevedevano questa possibilità. del Nord sono imprese di interesse strategico nazionale, signor Presidente. Siamo critici, perché la posizione del commissario Bondi riporta alla memoria la commedia del Goldoni «Arlecchino servitore di due padroni»: una cosa che probabilmente non è possibile. Critici perché l'evoluzione del caso Ilva sarà il banco di prova su cui verranno valutate le capacità di questo Paese di essere affidabile e coerente, non sempre abbiamo dato prova di questo nel passato, signor Presidente. Critici anche perché questa era l'occasione per riprendere, rafforzata, quella politica industriale che sembra L'Italia ha già 3 milioni di disoccupati, e di certo non bisogna fermare l'attività produttiva - questo la Lega Nord non l'ha mai chiesto perché fermare l'Ilva vuol dire conseguentemente mettere la parola fine alla siderurgia in Italia; perché fermare l'Ilva significa chiudere i siti di Genova Cornigliano, di Novi Ligure (che pure abbiamo visitato con le Commissioni) e di Racconigi.

Eppure l'area di Taranto, i suoi abitanti sono stati oggetto di quarant'anni di inattenzioni, di non opere, di omissioni. Probabilmente, signor Presidente, anche per mia colpa, ma sicuramente per vostra colpa, per vostra massima colpa. Le Commissioni attività produttive e ambiente hanno avuto modo di vedere da vicino la realtà degli stabilimenti di Taranto e di constatare la criticità della situazione per quanto attiene alla salute dei cittadini.

In una filanda di fine secolo, signor Presidente, ad una visita del re e della regina e dei figli del re, il proprietario aveva schierato in prima fila solo il personale presente in fabbrica: le ragazze più belle, gli uomini sani, i baldi giovanotti. Gli operai più malandati, i mutilati, gli ammalati, quelli che erano veramente storpi, li fece stare a casa. Ed è un po' quello che è successo durante la nostra visita all'Ilva, signor Presidente:

Non c'era fumo che uscisse da quelle ciminiere, non c'era un vento forte tipico delle zone di mare che portasse via i cumuli di prodotti residui delle fonderie che pure erano presenti nel plastico. L'obiettivo delle molteplici audizioni sia in Senato che in prefettura a Taranto e delle visite agli stabilimenti Ilva di Novi Ligure e di Taranto era quello era quello di costruire un quadro di informazioni e di conoscenze che tornasse utile nell'esame del decreto‑legge. Tutto questo lavoro, signor Presidente (glielo posso garantire), si è ridotto a un semplice arricchimento personale sulla questione del sito Ilva. Non sapevo nulla, adesso so tante cose.

Per questo motivo non abbiamo affatto sposato l'orientamento del «nulla modificare» volto ad evitare la decadenza del decreto. Signor Presidente, il «non toccare il macchinista» ha messo in condizione quest'Aula, la Camera alta, di avere in questo provvedimento un ruolo mai così basso un provvedimento che arriva in Senato e circa il quale si sa con certezza che nessuno avrà la possibilità di modificarlo. Signor Presidente, per l'attenzione che la Lega Nord ha avuto per questo decreto, per il lavoro che abbiamo svolto in Commissione,

come lui, signor Presidente, abbiamo avuto la certezza di fare un lavoro inutile; come Sisifo abbiamo spinto un masso su per la montagna per poi vederlo rotolare a valle. E per come vediamo le cose in quest'Aula siamo sicuri, signor Presidente, che questo non succederà per l'eternità, come accade per il povero Sisifo, ma solo sino alla fine di questa anomala legislatura sostenuta da un'anomala maggioranza.

Scelta Civica è favorevole al disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto Ilva. È un provvedimento che tenta di trovare un equilibrio avanzato fra problemi ambientali, di salute e di lavoro. Il testo inviato dalla Camera è - a nostro avviso - condivisibile, e la decisione di non presentare emendamenti - presa dei partiti di maggioranza su richiesta del Governo - viene, per così dire, attenuata dalla predisposizione dell'ordine del giorno G101, largamente condiviso, che impegna il Governo a intervenire tempestivamente su alcune tematiche emerse durante i lavori delle Commissioni in Senato, senza snaturare il decreto in oggetto. Il provvedimento individua nel commissariamento lo strumento più idoneo per superare le inottemperanze AIA in tempi prestabiliti e, nel contempo, garantisce che l'attività di impresa mantenga l'occupazione e generi quelle risorse indispensabili perché le inottemperanze AIA possano essere superate. Il provvedimento si preoccupa anche di garantire che la proprietà dello stabilimento - sospesa per una diversa e migliore gestione - sia comunque tutelata mediante provvedimenti di trasparenza e di garanzia, anche nella redazione del piano industriale. È importante sottolineare che, se da una parte viene soppressa la figura del Garante, dall'altra viene data al commissario un'ampia delega di comunicare alle comunità locali e al Parlamento quello che sta avvenendo all'interno dello stabilimento. Ed è anche importante che il provvedimento istituisca tre esperti sui tre punti critici di questa vicenda: la salute, l'ambiente e l'attività industriale. Vorrei concludere con due considerazioni di carattere più generale. Nella sua audizione presso le Commissioni ambiente ed attività produttive del Senato, il subcommissario Ronchi ha sottolineato il profondo significato etico della grandiosa operazione politica ed economica oggi in atto all'Ilva. Se un Paese manifatturiero come l'Italia, che consuma ogni anno quasi 30 milioni di tonnellate d'acciaio, rinunciasse a produrre buona parte dell'acciaio di cui ha bisogno, agirebbe in modo ecologicamente irresponsabile, scaricando su altri popoli i rischi ambientali e per la salute connessi a questo tipo di produzione. Dubito che nelle acciaierie dell'Ucraina - il primo Paese da cui l'Italia importa acciaio - siano rispettati rigorosi *standard* ambientali e di sicurezza del lavoro. Esistono fabbriche grandi come l'Ilva che riescono a produrre in modo ecologicamente sostenibile, come ad esempio la grande acciaieria di Duisburg in Germania. Dobbiamo accettare la sfida di farlo anche in Italia. Secondo Scelta Civica, le procedure identificate da questo disegno di legge e gli uomini a cui queste procedure sono state affidate sono una garanzia sufficiente per tentare di vincere la sfida. Infine, come sottolineerò assieme ad altri colleghi in un ordine del giorno che ci auguriamo il Governo accolga, la grande attenzione della politica su questi temi dovrebbe tradursi anche nella promozione, da parte del Governo, di studi più rigorosi sul rischio per la salute rappresentato dai grandi complessi industriali del passato e del presente. Gli studi oggi disponibili per l'Italia non utilizzano in modo intensivo i dati e le tecniche statistiche ed epidemiologiche oggi disponibili. È importante che questo *gap* venga rapidamente colmato, per garantire un monitoraggio sempre più rigoroso della salute dei cittadini e dei lavoratori. grazie.

rispettarlo nella forma, ma non nella sostanza. Allora, sostanzialmente, il provvedimento dice che qualunque stabilimento con un certo numero di dipendenti che venga dichiarato di interesse nazionale

se uno stabilimento viene commissariato, il commissario non è penalmente responsabile per quello che fa nell'attuazione dell'AIA per 36 mesi, né sono responsabili le persone che lui delega (quindi, può delegarne tantissime). Succede quindi che questo stabilimento opera in deroga ai principi dell'AIA, cioè può inquinare laddove qualcun altro che rispetta le prescrizioni dell'AIA non lo può fare: questa è una distorsione del mercato, perché qualcuno opera secondo regole

Lo ha detto lo stesso Bondi, definendole «siti temporanei di stoccaggio», che altro non sono che discariche a cielo aperto, che sono fatte senza il benché minimo controllo, tant'è che ci sono provvedimenti di sequestro della magistratura. Benissimo. nel momento in cui si concede al commissario di sistemare queste discariche a sua discrezione e non ne è penalmente responsabile, costui può stoccare rifiuti dalla composizione ignota, inquinare e non è penalmente responsabile, con ulteriore aggravio di costi per la collettività. Ovviamente l'Unione europea ci chiederà: ma perché permettete di fare questo? Seconda procedura d'infrazione. Terza possibile procedura d'infrazione (poi apriamo le scommesse). L'Unione europea potrebbe dire: c'è un commissario nominato dallo Stato, lo Stato sta aiutando qualcuno in favore di qualcun altro. E siamo a tre: aiuti di Stato. Tutte le volte siamo stati condannati su queste cose e non abbiamo ancora imparato. Qualcuno potrebbe dire: dopotutto abbiamo solo 104 procedure aperte, facciamo 107; cosa cambia per tre in più? Tanto siamo sempre noi a dover pagare. Questa è la verità: se vogliamo estendere il metodo Ilva e creare una selva di società commissariate che operano in deroga, diciamocelo. Personalmente

In conclusione, questo provvedimento fa acqua da tutte le parti. Ci sarebbe l'opportunità di lasciarlo andare, perché è un pessimo provvedimento, e mettersi d'accordo per farne uno migliore. Noi avremmo dato la disponibilità in Commissione a far sì che i nostri emendamenti contribuissero al miglioramento. Noi abbiamo sempre pensato che questo fosse il luogo in cui fare il miglior provvedimento di legge possibile e non quello di qualcuno o di qualcun altro: non esiste una legge di qualcuno! Le leggi sono di tutti: noi le approviamo, ma sono di tutti, e dovrebbe essere nostro preciso dovere fare il meglio che possiamo. Quando arriva qualcuno che ti dice, *gratis*:

E questo solo per l'area a caldo e per i parchi minerari. Non si parla assolutamente di bonifiche. Si chiama «autorizzazione integrata ambientale», ma non è questo: è autorizzazione integrata a mettere a posto lo stabilimento almeno un pochino. Questa è la verità: prendetela e fatene quello che volete. grazie. Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo,

Dall'altra l'ambiente, l'aria che respiriamo, l'aria che respiriamo io e i miei figli, i miei cari, l'aria, gli odori, la terra e il mare della mia provincia, della mia città e del mio territorio. Non posso, e come me non può nessuno dei miei colleghi del PdL pugliese, prescindere da alcuno dei due grandi temi che ruotano attorno l'*affaire* appunto, e ambiente. Da salvaguardare entrambi ovviamente. A molti - mi rendo conto - ciò potrà apparire utopistico; per me, invece, è assolutamente imprescindibile. Il futuro di Taranto e della nostra Regione, la Puglia, passa e passerà, oggi come tra un secolo, da una necessaria armonia di due facce della stessa medaglia chiamate ora a fondersi. Lo sappiamo noi senatori; lo sanno, ancor meglio di noi, le famiglie che chiedono alla Stato e al Governo il superamento di una fase giustamente ritenuta anacronistica. Questa, è la premessa che a molti, forse, apparirà solo ideologica perché i fatti, nel recente passato, hanno detto altro. irresponsabile anche solo ipotizzare la chiusura dello stabilimento, come se si trattasse di simulare con un programma informatico una casa senza fondamenta, senza tetto, persino senza porte. le ucronìe possibili di un territorio senza Ilva sono assolutamente inconcepibili per quanto radicato è tra gli altiforni un intero sistema occupazionale che lega a doppio filo professionisti, dipendenti, funzionari, operai e guardie giurate del territorio con azienda e stabilimento. La chiusura dello stabilimento, piuttosto, provocherebbe una frattura drammatica che non possiamo permetterci. Non possiamo farlo oggi, non potremmo farlo neanche domani se non saremo in grado di sviluppare nuove realtà imprenditoriali capaci di sopperire a ciò che l'Ilva, anno del Signore 2013, rappresenta per il sistema lavoro dell'intero Sud Italia, ma - aggiungerei - dell'intera Italia. La sfida, piuttosto, è e sarà un'altra: la vera sfida sarà quella di trovare soluzioni col tempo sempre più definitive che, consentendo allo stabilimento siderurgico più grande d'Europa di continuare a produrre, e quindi di non perdere ma, anzi, attirare nuovi investimenti, possano allo stesso tempo garantire le risorse indispensabili agli investimenti necessari per l'attuazione delle prescrizioni dell'AIA. occorre trovare soluzioni che con il tempo possano rendere - mi ripeto - lo stabilimento siderurgico più grande d'Europa anche il modello per eccellenza di un nuovo modo di fare industria in Italia, nella stessa Europa, nel mondo intero. L'Ilva, per oltre mezzo secolo, non ha prodotto bolle di sapone: questo ormai lo sappiamo tutti. Così come sappiamo che di errori nel passato ne sono stati commessi: dalla sua posizione, a ridosso della città e di un quartiere mortificato in virtù dello sviluppo del dio denaro, alle gravi, gravissime omissioni in tema ambientale. Ma l'Ilva ha anche rappresentato per intere comunità la speranza di una casa, dell'indipendenza economica, di un forse fittizio benessere per se stessi e per la propria famiglia. Tutela dell'ambiente e lavoro rappresentano diritti inalienabili per ogni singolo cittadino, per ogni essere umano. Per questo auspico che la discussione odierna sia mirata al tentativo intrinseco nel nostro mandato di migliorare, non di distruggere, di parlare di cose concrete che vanno, appunto, dall'aria che respiriamo e che respireremo alla busta paga del padre di famiglia o del giovane marito con ancora sogni e speranze. Il mio appello è rivolto al Governo, un Governo chiamato a mettere a disposizione risorse già stanziate per le bonifiche. Un Governo chiamato a monitorare con attenzione qualsiasi tipo di attività, *in primis* quelle finalizzate al rilascio dell'AIA. Un Governo che sappia analizzare, valutare e risolvere l'intero caso Taranto, dall'assenza e dalla carenza di infrastrutture alla crisi sociale. Un Governo che non metta i cittadini di fronte a una scelta impossibile: morire di fame o morire per l'aria che devono necessariamente respirare. grazie. il decreto-legge che ci accingiamo a convertire in legge introduce una novità profonda nell'esercizio dei diritti di proprietà ai fini della tutela dell'ambiente e della salute. Questo provvedimento prende le mosse da un'emergenza - quella dello stabilimento Ilva di Taranto - che rischia la chiusura per effetto del rifiuto dell'azionista di controllo, la famiglia Riva, di ottemperare pienamente all'autorizzazione integrata ambientale, emanata dal Ministero dell'ambiente: un rifiuto al quale la magistratura tarantina ha doverosamente reagito con provvedimenti restrittivi dell'attività aziendale. Questi provvedimenti, ove ove lasciati a se stessi, metterebbero a dura prova la continuità aziendale e, dunque, la continuità del lavoro. Se quindi è vero che questo provvedimento parte dall'emergenza Ilva, è anche vero però che esso apre una strada nuova per risolvere le emergenze ambientali andando oltre la dinamica tra azienda inadempiente e magistratura inquirente. Intendiamoci: la supervisione della procura e dei tribunali sul passato prossimo e sul passato remoto non può e non deve venir meno né oggi né mai, ma la costruzione del domani appartiene in primo luogo all'impresa e al complesso dei suoi *stakeholder*

quando questa rientri nell'elenco dei siti di interesse nazionale. In questi casi il Governo si assume la responsabilità di sospendere provvisoriamente i diritti della proprietà per ricomporre un equilibrio tra gli stessi diritti di proprietà e il diritto al lavoro e il diritto alla salute e alla vita in un ambiente che rispetti i parametri ecologici stabiliti su basi scientifiche, e dunque verificabili, dagli enti a ciò preposti (e non da quanto si è letto l'ultima volta cliccando su Google). L'istituzione del commissariamento è stata fin qui limitata ai casi di insolvenza da parte di imprese di grandi dimensioni e questo ha comportato la sparizione della vecchia proprietà, ormai incapace di far fronte agli obblighi con i creditori. Il caso Parmalat può essere assunto ad esempio sia per l'entità del dissesto, sia per l'esito felice del commissariamento, che ha consentito di recuperare oltre 2 miliardi dalle banche complici di Tanzi e di riportare al profitto l'azienda, salvando il grosso dei posti di lavoro. Nei casi di emergenza ambientale, invece, non sempre c'è insolvenza. Nel caso dell'Ilva, in particolare, lo stato patrimoniale appare ancora solido e i conti economici degli ultimi diciassette anni (mi sono preso la briga di andarmi a rileggere i bilanci) mostrano un margine operativo lordo cumulato di circa 7 miliardi di euro. Tuttavia la creazione di valore per gli azionisti è un obiettivo legittimo che trova il suo limite nel rispetto dei contratti, primi fra tutti quelli di lavoro, e nel rispetto delle leggi, prime fra tutte quelle ambientali. Per questo, la proprietà non viene cancellata, ma viene sospesa nell'esercizio dei suoi diritti per il tempo necessario - al massimo 36 mesi, recita il provvedimento - che si ritiene necessario per risanare l'ambiente degli stabilimenti. La scommessa che parte con questo decreto-legge è quella di risanare l'Ilva - e un domani le imprese che si trovassero nelle stesse condizioni - con i soldi generati dalla loro gestione per poi restituire alla proprietà un'azienda migliore, magari con qualche debito in più a causa degli investimenti ecologici, ma anche più efficiente e capace di riottenere presto equilibri più solidi. A questo scopo le Commissioni ambiente e industria del Senato hanno effettuato numerose audizioni e due importanti missioni a Taranto e a Novi Ligure, dove tutti sono stati ascoltati. A questo proposito mi piace ringraziare, per la solerzia e l'impegno profuso, i funzionari del Senato che ci hanno aiutato in queste missioni. Ebbene, le due Commissioni hanno presentato un ordine del giorno, accolto dal Governo, che intende rafforzare il commissario e il subcommissario su quattro fronti assai delicati (abbiamo presentato un ordine del giorno perché non era possibile, per le esigenze dei lavori parlamentari, fare diversamente). l'azienda commissariata ha bisogno di credito per investire; poi, lavorando, rimborserà ma all'inizio, senza la fiducia delle banche, non parte. Per questo ci vuole la prededucibilità dei nuovi finanziamenti in caso di *default* (parlo dei nuovi finanziamenti per il commissariamento, non dei vecchi che seguono il corso normale). In secondo luogo, il commissario deve poter risolvere ed eventualmente rinegoziare i rapporti con le parti correlate (nel caso specifico, così tutti ci capiamo, con le società appartenenti al gruppo Riva ma non al gruppo Ilva). È tipico delle aziende come l'Ilva, che fanno parte di gruppi più grandi, delegare alle *holding* di controllo tutta una serie di funzioni e di informazioni che significano soldi e potere. Bondi o non Bondi, se Riva conserva il controllo dei sistemi informatici e della tesoreria nessun commissario potrà mai andare lontano. In terzo luogo, commissario, subcommissario e i tecnici da loro delegati vanno protetti dalla responsabilità oggettiva, sancita dalla legge n. nel momento in cui entrano a lavorare su una scena che, al momento, non rispetta la legge; diversamente nessuno potrà fare questo lavoro. Stiamo lavorando per risanare e rimettere in riga l'azienda; è evidente che all'inizio non lo è. Quarto punto. La gestione dei rifiuti, sia di quelli ereditati sia di quelli che saranno prodotti lavorando, va ricondotta a normalità, attraverso l'intervento del Ministero dell'ambiente su proposta del commissario e sentite la Regione e Ci auguriamo che questi punti, necessari al buon svolgimento dell'opera del commissario e del subcommissario, vengano accolti dal Governo nel primo provvedimento utile. Senza un commissariamento forte e trasparente, obbligato a rendere conto al Parlamento e ai territori, ma al tempo stesso non dimezzato da assemblearismi rissosi e dunque, proprio in quanto non dimezzato, pienamente responsabile, il rischio per l'Ilva e le aziende che si troveranno nelle stesse situazioni è la morte per asfissia. C'è tutto un mondo che non vuole l'Ilva risanata, ma la vuole morta. Anzitutto i concorrenti europei ed extraeuropei, ai quali non parrebbe vero vedere sparire altiforni che erano e restano tra i più produttivi del vecchio continente. E non parrebbe vero a loro evitare di avere un *benchmark* che li costringerebbe a una rincorsa sul piano degli investimenti ambientali. Ma poi c'è tutto un mondo che sogna la sostituzione del reddito produttivo, fatto nel rispetto dell'ambiente e della salute (lo vogliamo ripetere ancora una volta), con i sussidi pubblici: sussidi per la disoccupazione, che si renderebbero inevitabili nel caso saltassero i 16.000 posti di lavoro connessi all'Ilva di Taranto, e sussidi per la bonifica di quell'enorme sito industriale, perché - ricordiamocelo - se l'Ilva chiude i Riva lasceranno fallire la società e la bonifica sarà posta a carico delle finanze pubbliche, non certo private. un'opera senza fine, a spese dello Stato come sarebbe la bonifica di un'Ilva chiusa, costituirebbe anche il terreno più adatto alle infiltrazioni del crimine organizzato, alle mafie degli appalti: diciamocelo oggi, per non doverci stupire poi domani e gridare allo scandalo. In conclusione, un'ultima osservazione. Oggi l'Occidente sta riscoprendo l'importanza dell'industria. Aveva creduto, sull'onda della globalizzazione finanziaria, che le banche, le borse valori, i commerci e i servizi fossero sufficienti a tenere in piedi le società avanzate. La grande crisi dalla quale non siamo ancora usciti ci ha rivelato che quel tipo di globalizzazione, che unifica tutto ma non i diritti e meno che mai i diritti del lavoro, ha generato regresso e impoverimento per la maggioranza delle persone che vivono del proprio lavoro. La ripresa, dall'America democratica di Obama al Regno Unito del conservatore Cameron, dal Giappone alla Germania, passa attraverso il rilancio dell'industria, non attraverso il rilancio delle parole. Salvare l'Ilva salvando l'ambiente è una scommessa da vincere per tutti noi. Spacciare la deindustrializzazione oggi della Puglia, domani dell'Italia come un successo ambientalista, invece, equivale a rendere un servizio non retribuito così immagino - al capitalismo finanziario che non elimina l'acciaio e neppure ama l'ambiente, ma preferisce una siderurgia lontana e non importa se, laddove finirà, inquinerà ancor più di oggi il nostro pianeta.

danno il senso della comprensione piena dello sforzo che stiamo compiendo tutti per affrontare una situazione unica nella storia industriale del nostro Paese. Una situazione che riguarda innanzitutto una grande città del Mezzogiorno, che vive un dramma nel conflitto che è esploso tra il lavoro, l'ambiente e la salute. Una situazione di straordinaria difficoltà del più grande impianto siderurgico d'Europa e degli oltre 15.000 lavoratori diretti e indiretti che vi trovano lavoro, un pezzo decisivo del futuro industriale del nostro Paese nella competizione internazionale. Quindi, il dibattito sicuramente ha colto in grandissima parte - ripeto - il senso vero delle questioni che sono alla base anche di questo ulteriore provvedimento al nostro esame. ribadire un concetto, che pure è emerso nel corso della discussione: non siamo di fronte ad un calcolo meramente burocratico di natura opportunistica nel momento in cui la maggioranza dei Gruppi decide di affrontare con responsabilità la necessità di convertire questo decreto in legge per evitarne la decadenza, che rischierebbe di verificarsi nel momento in cui dovessimo immaginare un ulteriore passaggio alla Camera dei deputati. Abbiamo deciso consapevolmente di portare a compimento l'*iter* di questo decreto perché non osiamo immaginare cosa potrebbe comportare la decadenza di un provvedimento al cui interno vi sono scelte che molti di noi ritengono e il Governo ha ritenuto decisive per l'obiettivo di salvare insieme il futuro industriale di quello stabilimento, l'occupazione, la tutela della salute, lo sforzo di risanamento ambientale della città e dello stabilimento dell'Ilva di Taranto. La decadenza del provvedimento comporterebbe il venir meno del commissario straordinario e, quindi, la riconsegna - lo richiamava per ultimo il collega Mucchetti - alla alla proprietà della gestione di quello stabilimento, a quella proprietà che si è resa responsabile in questi anni non solo di clamorose clamorose violazioni della tutela ambientale sanzionate dall'intervento della magistratura, ma che ha mostrato totale irresponsabilità negli ultimi mesi non adempiendo neppure alle prescrizioni stringenti dell'autorizzazione integrata Verrebbe meno, in secondo luogo, l'obbligo a redigere, all'interno del procedimento dell'AIA, il piano delle misure per la tutela dell'ambiente e della salute e contemporaneamente il piano industriale, piani programmatori di interventi funzionali alla piena applicazione dell'AIA. Verrebbe meno, ancora, il vincolo, che questo provvedimento definisce in maniera inequivoca, di destinare tutte le risorse rivenienti dalla continuità produttiva dello stabilimento Ilva di Taranto prioritariamente al risanamento ambientale e all'attuazione delle prescrizioni dell'AIA. Verrebbe meno inoltre rivolgo questo riferimento in particolare alla collega De Petris, con cui abbiamo molto ragionato in questi giorni, seppure con opinioni diverse

Verrebbe meno, infine, lo sblocco di una parte delle risorse definite un anno fa con un protocollo d'intesa recuperato nel decreto-legge dello scorso agosto, con cui si destinano risorse all'attività di bonifica. Ecco, questo è quello che verrebbe meno

i compiti precedentemente assegnati al Garante per l'AIA, si adoperino perché ci sia un colloquio costante in termini di informazione, di ascolto, di consultazione con le comunità locali. Penso che questo compito, attribuito al commissario, dottor Enrico Bondi, debba essere svolto

Un clima sociale in cui tutti i soggetti, dalla cittadinanza attiva alle forze sociali e sindacali, alle istituzioni locali, agli enti ispettivi, a chi oggi ha il compito di gestire l'azienda in questo passaggio così delicato, si ascoltano reciprocamente per costruire una sintesi sostenibile non è un fattore indipendente per la buona riuscita di questo straordinario ed unico tentativo di mettere in campo un'operazione che salvi l'azienda e i posti di lavoro, ma avvii contemporaneamente una grande opera di risanamento ambientale e di tutela della salute. Di tutto ciò sono consapevoli, credo, sia il commissario che il Parlamento. Tutti noi vigileremo insieme al Governo grazie.

una parte degli elementi di criticità che è stata ribadita in alcuni interventi attiene alla mancanza di criteri per la nomina.

non hanno considerato che qui ci troviamo di fronte ad una fattispecie totalmente diversa che necessitava di una figura di per sé ancora più straordinaria di quella che normalmente è implicita nel concetto stesso di commissario. Il commissario acquisisce - si è detto - anche i poteri che aveva il Garante nei precedenti interventi fatti dal legislatore e, in particolare, nei decreti anno. La figura del Garante, di per sé, aveva una sua funzione e una sua validità, ma poi l'attività realmente svolta, per quello che abbiamo potuto constatare, non è stata così copiosa e così significativa, per cui può essere tranquillamente, non dico surrogata, ma ricompresa nei poteri, nei compiti e nelle mansioni che verranno affidate al commissario,

ma che, con gli strumenti attuali di partecipazione e di condivisione che si possono individuare, possono essere compiti tranquillamente affidati al commissario.

la discussione viene influenzata continuamente dalla vicenda di Taranto. Qui le esigenze della produzione sono quelle di una città in crisi e non solo per l'Ilva, perché essa non ha più quel significativo insediamento di attività militari che aveva nell'Italia del dopoguerra. L'Ilva rimane comunque lo stabilimento di un'azienda importante per quel tipo di città. Fra l'altro, c'è il rischio che, con scelte non strategiche (richiamo qui l'intervento del presidente Mucchetti), l'Italia si allontani definitivamente dal mercato dell'acciaio e risolva, per esempio (è stato detto in interventi delle scorse settimane), il problema della sovrapproduzione europea dell'acciaio, implicitamente eliminando solo se stessa, ma risolvendo il problema della sovrapproduzione europea. Questa sarebbe una beffa non per Taranto, ma per il sistema italiano.

Dobbiamo dire una cosa importante: il progetto Sentieri, che è stato più volte richiamato, e tutte le indagini epidemiologiche dividono notevolmente la comunità scientifica e evidenziano quanto sia necessaria una nuova attività di ricerca e di epidemiologia che possa portare a dati molto più univoci ed oggettivi, che consentano una più facile lettura del problema.

con articoli diversi che qui è inutile ribadire, trovano comunque la sintesi in questo decreto che, di fatto, è figlio dell'articolo 41 della Costituzione:

nuova finestra"). La Presidenza, conformemente a quanto già stabilito dalle Commissioni riunite in sede referente, dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, l'emendamento 2-*ter*.0.1 relativo al pagamento dei debiti delle Province, in quanto estraneo all'oggetto della discussione. Dichiara altresì inammissibile, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento, l'emendamento 1.56, in quanto privo di portata modificativa.

1a Commissione permanente, esaminati il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni: - in merito all'articolo 2-*bis*, si rileva che le risorse utilizzate a copertura, a valere sul Fondo per esigenze di tutela ambientale, rivestono natura di conto capitale e, tuttavia, sono stornate per un intervento che, sia pure di portata limitata (90.000 euro per ciascuno degli anni del

si segnala che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione dei contributi pluriennali, ivi utilizzato a copertura, dovrebbe essere esclusivamente finalizzato a compensare gli effetti negativi, in termini di cassa, scaturenti da specifici contributi di importo fisso costante, con oneri a carico dello Stato,

da una clausola di neutralità finanziaria, la Convenzione internazionale richiamata dal dispositivo prescrive una serie di adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche in materia di informazioni ambientali, con il rischio di vanificare la predetta clausola di neutralità finanziaria».

Grazie

Il provvedimento si occupa del sito di interesse strategico nazionale in Italia esistono altri 56 SIN meritevoli di altrettanta considerazione. Con il nostro ordine del giorno G100 chiediamo al Governo di impegnarsi a definire, assieme alle Regioni, un piano nazionale per le bonifiche dei SIN contenente impegni finanziari certi e procedure di semplificazione atte ad avviare l'attività di ripristino ambientale. Per quanto riguarda invece l'ordine del giorno G103, tenuto conto che il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire non risolve affatto il problema cogente dello smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, nonostante all'interno della fabbrica di Taranto esistano due discariche che hanno avuto il via libera della valutazione d'impatto ambientale, (nonostante ci sia stato negato l'emendamento) di impegnare il Governo ad adottare tutte le iniziative affinché nel più breve tempo possibile queste due discariche vengano vengano autorizzate. Segnalo all'Assemblea che lo smaltimento dei rifiuti nell'attività industriale e dei materiali di bonifica comporta una spesa valutata dal subcommissario di 300 milioni di euro.

che permettano di avanzare in modo significativo la ricerca di connessioni tra causa ed effetto nel legame tra malattie e rischi ambientali.

didefinire, in raccordo con la Regione competente, tempi e modalità per la messa a norma delle discariche di cui in premessa, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria ed al fine di garantire il massimo grado di protezione dell'ambiente.

a capire come mai il relatore e il Governo hanno espresso un parere contrario sull'ordine del giorno G103. Peraltro, l'aspetto delle discariche è uno degli ambiti oggetto di delega al Governo nell'ordine del giorno della maggioranza approvato

questo apre la strada al conferimento in discarica di materiali dalla composizione non stabilita, nel senso che per stessa dichiarazione del commissario del commissario non c'è la classificazione merceologica di questi prodotti. Quindi, rischiamo che vadano in discarica delle cose che sono autodichiarate essere pericolose o non pericolose, e questo non può essere assolutamente

così come quella delle acque, debba essere ricompresa all'interno delle procedure dell'AIA stessa, e non con un decreto a parte o con una specie di sanatoria. La questione è molto delicata: noi dobbiamo evitare - questo varrà anche per altre questioni - che il commissariamento ai fini ambientali possa produrre grazie. replicato, a tenere in grande considerazione queste valutazioni, perché introdurre, così come prevede l'ordine del giorno della maggioranza, la questione delle discariche nel primo decreto che passa esporrà ancora una volta il nostro Paese, per quella situazione, ad una procedura di infrazione.

Mi dispiace, ma il vostro tempo contingentato è già scaduto, quindi noi possiamo accettare solo le dichiarazioni Interverrà sul prossimo.

Per quanto riguarda invece l'ordine del giorno G105, impegniamo il Governo ad adottare opportune iniziative affinché i rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti dalle bonifiche del SIN di Taranto siano smaltiti all'interno del medesimo territorio regionale.

ma esclusivamente lo stabilimento di Taranto, visto che i tre stabilimenti allocati al Nord, quelli di Genova, Novi Ligure e Racconigi, non hanno problemi di inadempienza con l'AIA.

che effettivamente possa sussistere un conflitto di interessi visto che si è andati a nominare quale commissario straordinario dell'impresa Ilva una persona che, seppur per un breve periodo, di amministratore delegato della stessa e quindi è certamente corresponsabile degli inadempimenti delle prescrizioni dell'AIA che hanno determinato poi l'intervento della magistratura.

per quanto riguarda la valutazione del danno sanitario il rapporto del danno sanitario deve legittimare la Regione competente a chiedere immediatamente il riesame

prevede che per commissariare un'azienda l'inosservanza in tema ambientale debba essere reiterata.

coinvolgere rispettivamente il Ministro della salute e le Commissioni parlamentari competenti nella scelta del commissario che il parere delle Commissioni sia anche vincolante. il Ministro della salute sia sempre presente nelle decisioni. L'emendamento 1.202 invece fa riferimento ai criteri di professionalità e di compatibilità meglio dire, di incompatibilità

grazie.

andasse a modificare le prescrizioni dell'AIA anche in corso. Il rapporto di valutazione di danno sanitario annuale deve essere condizione di modifica dell'AIA. Ancora, con l'emendamento 1.72 chiediamo di sopprimere il comma 9,

Presidente, l'emendamento 1.14 è molto semplice da illustrare: praticamente chi svolge il ruolo di commissario sicuramente deve essere una persona terza; abbiamo

Prego,

si attua nella conservazione della continuità aziendale. Noi vorremmo che si aggiungessero le parole: «nonché alla salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale e di rispetto di adeguati parametri di tutela sanitaria»,

Presidente, l'emendamento 1.214 mira alla cancellazione della parte del comma 7 dell'articolo 1 in cui si prevede che i rapporti di valutazione del danno sanitario prescritti dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, debbano conformarsi ai criteri metodologici fissati dal decreto-legge oggi in discussione. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può modificare unilateralmente le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale ma legittima la Regione a richiederne il riesame. Orbene, è evidente che qualora il suddetto comma 7 dell'articolo 1 fosse approvato nella sua attuale formulazione, come licenziato dalla Camera dei deputati, verrebbe del tutto eliminato il senso della valutazione del danno sanitario, ossia l'unico strumento in grado di misurare le ricadute sul piano sanitario dell'Ilva di Taranto e di indicare, sulla base dei risultati ottenuti, eventuali ulteriori prescrizioni a difesa dell'ambiente e della salute.

L'emendamento 1.209 è volto ad assicurare il diritto alla trasparenza perché noi riteniamo che, attraverso la pubblicazione dei dati sul sito *web* del Comune sia la proprietà sia, a maggior ragione, i cittadini che vivono nell'area dello stabilimento interessato possano avere informazioni in tempo reale sull'andamento della situazione sanitaria e soprattutto sulla gestione di tutto impianto. Il fine è quello di garantire il diritto alla salute e il diritto alla conoscenza di chi vive queste drammatiche situazioni.

Mi scuso con i colleghi senatori se stiamo perdendo qualche minuto, però, sempre citando l'articolo 109 del Regolamento di quest'Aula, al comma 2 si legge: «Fatta quest'Aula, al comma 2 si legge: «Fatta eccezione per i casi in cui il Regolamento prescrive la esclusione o la limitazione della discussione, un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare

in cui il Regolamento prescrive l'esclusione o la limitazione», dato che il tempo contingentato è già terminato. È stata già affrontata stamattina questa posizione. Passiamo alla votazione

Passiamo alla votazione della

Signor Presidente, mi sembra che la notazione del collega Martelli, assolutamente logica ed ineccepibile, non abbia ancora avuto risposta. Quindi, volevo sollevare la questione in quanto, a nostro avviso, si potrebbe anche leggere il Regolamento in quel modo dando voce al dissenso, posto che sia possibile capire quale sia la volontà del Gruppo. Ma se non è possibile esprimere questa volontà, neanche il dissenso potrà essere espresso.

Passiamo alla votazione

senatore Santangelo).* Vorrei cercare di evitare di rallentare i lavori per queste motivazioni, invitando soprattutto al massimo della correttezza del comportamento da parte di tutti coloro che sono ai loro posti e diligentemente procedono alla votazione nella loro postazione, evitando di essere fuori posto nel momento della votazione o di incaricare qualcuno di votare al proprio posto. Prego

a fronte di reiterati comportamenti che violano lo spirito della norma. La preghiamo pertanto di far rispettare, anche e soprattutto per questi casi,

votazioni e io sono rimasta in piedi, senza le che lei si sia minimamente degnato di darmi la parola. Adesso dichiaro il voto favorevole all'emendamento 1.41.

che prevede una esenzione dai *ticket* sanitari per tutte quelle persone che vivono nei pressi delle aree soggette all'inquinamento.

Ricordo che nel decreto approvato è previsto che le Regioni dovessero presentare entro il 15 maggio di quest'anno i relativi programmi in attuazione della legge per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari.

di piccole residenze sociosanitarie inserite nei contesti sociali e anche i relativi programmi riabilitativi. Inoltre, sembra che non sia rispettato il potenziamento dei servizi di salute mentale dei territori e che le proposte e che le proposte fatte debbano escludere la riproduzione di soluzioni manicomiali, magari più eleganti nella loro strutturazione, ma che di fatto replicherebbero i manicomi. Grazie, non possiamo e non dobbiamo permettere che la legge non sia applicata. Non possiamo tornare ancora una volta ad un nuovo rinvio, com'è stato fatto d'altra parte quest'anno. Pur conoscendo le difficoltà dei territori ritengo che

civiltà, di rispetto, ma anche, sostanzialmente, per questo Parlamento e questo Governo, una risposta di efficienza e di efficacia delle istituzioni. Chiedo quindi una risposta, perché il silenzio e il ritardo del Governo creano qualche preoccupazione.

lo scempio ambientale che si sta verificando nella zona collocata tra le vie Laurentina e Castel di Leva, a danno del complesso monumentale medievale di Tor Chiesaccia, risalente al X secolo d.C. e sottoposto a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nonostante sia vincolata all'inedificabilità dal piano paesaggistico della Regione Lazio n. 15/3 l'area intorno alle rovine di Tor Chiesaccia è oggetto di innumerevoli violazioni e difformità urbanistiche a causa di alcune concessioni edilizie, allegramente assegnate al gruppo imprenditoriale Caltagirone. Permessi che hanno tranquillamente consentito la costruzione di palazzi molto più alti, fino a 5 piani in più, rispetto alle prescrizioni contenute nella valutazione d'impatto ambientale regionale, dove l'area risulta destinata a verde e servizi pubblici. Tali costruzioni, oltre a essere innalzate sulle mura del campo fortificato e una necropoli, derogano spudoratamente al divieto di edificare o alterare i terreni entro i 100 metri dalla Torre, come stabilito in un decreto della Direzione regionale della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, che vieta inoltre di «precludere con eventuali costruzioni il profilo e la percezione della Torre», preclusione inevitabile se due palazzoni di sette piani fossero edificati. A ciò si aggiungono il proliferare di incendi dolosi volti a danneggiare i monumenti e il crollo, verificatosi nel gennaio scorso, di una parte della chiesa medievale (qui si parla spesso di tutelare e non tuteliamo) a causa delle vibrazioni prodotte da escavatori e camion operanti nel cantiere. PRESIDENTE. Presidente, concludo. Chiedo, pertanto, in quest'Aula un intervento decisivo del Governo e del Ministro per i beni e le attività culturali affinché sospenda tutte le concessioni rilasciate dal Comune di Roma, in quanto l'area - come si legge in una relazione dello stesso Ministero di qualche anno fa - «si distingue per l'alta qualità paesaggistica, l'ampiezza dei quadri panoramici, la stratificata articolazione del sistema insediativo storico notevole diffusione di beni archeologici e architettonici». È urgente verificare per quale motivo l'istruttoria prodotta dal responsabile di zona

Presidente, deluderò il collega Scibona ma, siccome sono giornate di grande lavoro, la volevo ringraziare personalmente per la conduzione dell'Aula di quest'oggi. È il suo lavoro e il suo mestiere, ma ogni tanto va riconosciuto che in situazioni difficili

Presidente, intervengo solo per fare una segnalazione. Poiché venerdì prossimo, il 2 agosto, cade l'anniversario della strage di Bologna, noi ci permettevamo di fare questa segnalazione per togliere il Consiglio di Presidenza dall'imbarazzo in cui si è trovato già il 27 giugno, per la commemorazione della strage di Ustica. Vorremmo allora aiutarlo a ricordarsi di chiedere di osservare un minuto di silenzio in memoria di queste vittime. Grazie.

Signor Presidente, intervengo a titolo personale in riferimento a questa mattina, quando ho ritenuto di dover lasciare l'Aula. Il problema è in ordine all'applicazione ed all'interpretazione del Regolamento ed eventualmente anche a ciò che era stato chiesto dal presidente Zanda in riferimento all'eventualità di demandare alla Giunta per il Regolamento. Io credo che il Regolamento, essendo uno strumento normativo paracostituzionale,

questo sarebbe un modo surrettizio di modificare il Regolamento. mi è stata tolta la parola. Ricordo che l'articolo 92 al comma 1 prevede che: «I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorità di una discussione o votazione hanno la precedenza

intervengo, come altri colleghi prima di me hanno fatto, in merito alla revisione della geografia giudiziaria, argomento sul quale ho presentato un'interpellanza relativa a Castelvetrano in data 20 giugno 2013.

è atteso in Aula dalla stragrande maggioranza dei senatori. Le chiedo in questo breve intervento di mettere in moto tutte le procedure necessarie alla calendarizzazione nel più breve tempo possibile di questo disegno di legge che risulta essere urgente, considerato che il 13 settembre entrerà in vigore la riforma.

il che significa che o non c'è l'impianto di aspirazione, oppure non è sufficientemente dimensionato, oppure è temporaneamente guasto. Le chiedo di trovare una soluzione definitiva, ma nel frattempo di trovare una soluzione temporanea che possa evitare che il fumo si sparga nei corridoi e, quando ci sono le porte aperte, entri anche in quest'Aula.

lei sa, la sala era adibita ai senatori per il decoro del Senato e dei senatori stessi. Ultimamente, ancorché nobile, è stata cambiata la sua destinazione d'uso ed è stata messa a disposizione per rilasciare interviste. Io credo che debba essere ripristinato l'uso precedente proprio perché al Senato afferiscono associazioni, cittadini, comitati che si incontrano con singoli

lungo i corridoi o sedute nella Sala Garibaldi o nella Sala Mazzini, ovviamente quasi uno sopra l'altro, uno addosso all'altro. Non è un bel vedere. Credo che queste associazioni, questi comitati meritino di essere ricevuti dai colleghi senatori in una sala che rispetti il decoro

mi è stato riportato - poi l'ho letto nel Resoconto stenografico della seduta odierna - che la senatrice Lezzi del Gruppo Movimento 5 Stelle, nell'intervento svolto oggi pomeriggio, oltre ad insultare il Partito Democratico e pressoché l'intera Assemblea, ha fatto il mio nome

grave soprattutto che la senatrice Lezzi, approfittando della mia assenza dovuta al fatto che ero impegnato nel lavoro di Commissione per la preparazione della conversione di un decreto-legge, si sia permessa affermazioni